Dopo l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri avrà luogo la discussione, i cui tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi per complessive due ore, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo. Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri, professor Conte. Signor Presidente, gentili senatrici e gentili senatori, il prossimo Consiglio europeo sarà il terzo al quale partecipo da quando ho l'onore di presiedere il Governo. Tradizionalmente il Consiglio europeo di dicembre ambisce, come ultimo appuntamento dell'anno del massimo organo rappresentativo dei Governi dell'Unione europea, a segnali chiari e oserei dire anche a decisioni significative sui temi prioritari dell'agenda europea. Questo Consiglio europeo assume una particolare valenza politica, giacché esso si svolge cinque mesi prima delle elezioni per il nuovo Parlamento europeo. La legislatura europea è dunque giunta al suo ultimo tratto, il che evidentemente restringe la possibilità di tradurre le decisioni in un *iter* completo con l'attuale Parlamento europeo e con l'attuale Commissione europea. Il Consiglio europeo affronterà anche il tema della Brexit, con una discussione a 27, dopo il rinvio del voto di ratifica dell'accordo di recesso da parte britannica, che, come sapete, era previsto per quest'oggi. Dopo il dibattito alla Camera dei comuni, il Governo britannico chiede maggiori rassicurazioni sul fatto che la questione irlandese sarà risolta nell'ambito delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito e che non entri in vigore la soluzione di riserva che, come noto, è prevista dal protocollo dell'accordo di recesso, il cosiddetto *backstop*, concordato dai negoziatori dell'Unione europea e britannici lo scorso novembre. Discuteremo

del *premier* britannico Theresa May. Guardiamo con profondo rispetto al dibattito democratico che si sta svolgendo a Londra, ma nello stesso tempo, a poco più di tre mesi dalla data fissata per la Brexit, dobbiamo sottolineare l'esigenza che l'uscita del Regno Unito dall'Unione avvenga in maniera ordinata, nell'interesse di fornire certezza e chiarezza ai tanti cittadini, tra cui molti italiani, e alle tante imprese, che sono coinvolti in questo processo. In un contesto che contiene ancora elementi di incertezza, continueremo pertanto a lavorare con i *partner* europei e con le istituzioni dell'Unione per prepararci anche allo scenario, per noi poco auspicabile, di un recesso senza accordo. L'avvicinarsi della fine della legislatura europea vede anche una crescente influenza sulla capacità decisionale del Consiglio dell'improcrastinabile esigenza di misurarsi col sempre più vicino bilancio politico che i cittadini europei tracceranno con il loro voto che, come sapete, è calendarizzato per la fine del mese di maggio 2019. Al Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre, pertanto, si dovrà tenere in debita considerazione direi il più ampio orizzonte politico di un'Europa in evoluzione in una fase di transizione; un'Europa di cui fra poco più di tre mesi il Regno Unito non sarà più membro; un'Europa in cui è sempre più chiara e urgente l'aspettativa dei cittadini di poter contare su istituzioni europee e nazionali che garantiscano maggiore equità, crescita, lavoro e sicurezza a tutto il nostro Continente. È dunque con un approccio ispirato al principio di responsabilità, sia verso coloro che ci hanno eletto sia verso le future generazioni, che perseguiamo l'obiettivo di un'Europa più equa e più sicura; e ci adopereremo in tale direzione anche in questo finale di legislatura europea. La priorità ineludibile di lavorare oggi per un futuro migliore dell'Europa è il filo conduttore dei principali temi che sono in agenda al prossimo Consiglio europeo: la gestione europea dei flussi migratori, in attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo dello scorso mese di giugno; l'impulso al negoziato per nuovo bilancio europeo pluriennale (il cosiddetto quadro finanziario pluriennale); e le prospettive della riforma dell'unione economica e monetaria. Per la discussione all'Eurosummit vale una considerazione che si applica anche al nostro rapporto con l'Europa con riguardo alla legge di bilancio. Occorre infatti superare un rigorismo miope che pretende di combattere l'instabilità con misure che invece finiscono per favorirla. Nel far avanzare l'unione bancaria e l'unione monetaria ed economica, l'Europa deve perseguire un rapporto finalmente equilibrato tra riduzione e condivisione del rischio. Considero inoltre essenziale che l'Eurosummit possa avviare una discussione realistica nei prossimi mesi sul bilancio dell'eurozona. È ormai evidente, specie dopo la crisi finanziaria, l'esigenza di affiancare gli strumenti accentrati di politica monetaria con una leva fiscale ugualmente centralizzata, che permetta di attenuare le tendenze alla divergenza e gli effetti di possibili *shock* asimmetrici. L'eurogruppo il 4 dicembre ha visto purtroppo confermata, nell'esaminare la proposta franco-tedesca al riguardo, la netta distanza tra gli Stati membri. In particolare, se da un lato si è registrata una disponibilità ad approfondire la possibilità di istituire un bilancio comune per le finalità di convergenza e di aumento di competitività, dall'altro lato permane un forte contrasto di vedute sull'ipotesi di attribuire al bilancio comune anche la funzione di stabilizzazione. Quindi l'avanzamento di questo progetto va valutato con cautela riservando una particolare attenzione a tutti i profili e i passaggi che lo caratterizzano. Quanto al completamento dell'unione bancaria, la nostra visione richiede che la riduzione del rischio sia finalmente accompagnata da corrispondenti misure di mutualizzazione dello stesso. Comprendiamo che sia ritenuto ineludibile un differente *timing* su due aspetti; apprezziamo che si proceda con l'istituzione di una misura di condivisione del rischio, quale sarà il *common backstop* per il Fondo di risoluzione unico. Pur tuttavia, il nuovo rinvio delle decisioni sullo schema assicurativo sui depositi è per noi il segnale di un'Europa che continua a farsi condizionare dai mercati piuttosto che tentare di indirizzarli. Quanto alla riforma della *governance* del meccanismo europeo di stabilità, manteniamo le nostre riserve su un approccio intergovernativo ribadiamo che i ruoli attribuiti al meccanismo europeo di stabilità non devono minare irreversibilmente le prerogative della Commissione europea, in particolare in materia di sorveglianza fiscale. Per quanto riguarda il tema della migrazione, il Consiglio europeo dovrà esaminare i prossimi passi, volti a compiere finalmente progressi concreti nell'attuazione delle conclusioni del giugno scorso. Il testo delle conclusioni indica che il Consiglio affronterà il *comprehensive approach to migration*. In questa sede intendo ribadire ai colleghi europei che è ora di far seguire finalmente alle parole i fatti e di dare corpo ad una regolazione e gestione dei flussi migratori che sia di matrice autenticamente europea. Per essere tale, essa non può più eludere la sfida prioritaria dei movimenti primari e della gestione dei salvati in mare. In particolare, non può più gravare sui Paesi di primo arrivo l'onere legato alla gestione degli sbarchi ed occorre - lo rivendico dall'estate - un coordinamento europeo fin dalla fase di sbarco. Un meccanismo di gestione dei salvati in mare richiede, inoltre, uno sforzo condiviso e azioni congiunte, proprio per aderire alle conclusioni del Consiglio europeo di giugno, in tre (le riassumo) componenti fondamentali: lo sbarco, che deve vedere uno sforzo condiviso degli Stati membri, col coordinamento, ovviamente, della Commissione europea. In secondo luogo, su cui ribadirò la necessità ineluttabile che gli Stati membri (e non solo quelli costieri e pertanto di primo arrivo) si facciano carico di uno sforzo realmente condiviso. Non posso accettare quanto propongono alcuni Stati membri, ossia la limitazione della redistribuzione dei salvati in mare alla sola categoria degli aventi diritto alla protezione internazionale; una simile opzione implicherebbe, peraltro, un onere aggiuntivo sui Paesi di sbarco, complicando l'efficace gestione europea degli sbarcati, anziché semplificandola, come sostengono gli Stati membri preoccupati quasi esclusivamente dei movimenti secondari. Terzo aspetto, anch'esso fondamentale, riguarda i rimpatri dei salvati in mare non aventi diritto alla protezione internazionale. Occorre che si dia finalmente sostanza a una europeizzazione dei rimpatri, ad esempio attraverso il mutuo riconoscimento, almeno negli Stati membri che vorranno procedere in questa direzione, delle decisioni in materia ed attraverso l'utilizzo della cooperazione allo sviluppo come incentivo per una migliore cooperazione con i Paesi terzi. Dico questo nella prospettiva di quell'investimento, *in primis* di stabilizzazione politica e di impulso alla crescita, che reputo indispensabile nei confronti dell'Africa, un Continente verso il quale l'Italia mostra particolare attenzione, come anche testimoniato di recente dalle mie visite in Etiopia, Eritrea, Algeria e Tunisia. Nella stessa direzione va l'impegno italiano ed europeo per la stabilizzazione e lo sviluppo della sponda Sud del Mediterraneo allargato, regione segnata da crisi umanitarie, recenti conflitti, ma anche terra di grandi opportunità, la cui realizzazione in termini di sicurezza e prosperità è nostro comune interesse promuovere. Sempre in tema di migrazione, ricorderò ai colleghi europei che l'Italia considera inaccettabile, perché irrealistico nella sua effettiva attuazione, lo spacchettamento della riforma del sistema europeo comune di asilo. Senza la riforma del Regolamento di Dublino, approvare gli strumenti legislativi del sistema già avanzati costituirebbe un *vulnus* politico alla logica del consenso e sarebbe, al contempo, controproducente sul piano tecnico, proprio per il nesso tra i predetti strumenti e il Regolamento di Dublino. Consideriamo inoltre essenziale che ci sia finalmente adeguata attenzione alla dimensione esterna, anche sul piano finanziario. Il *trust fund* per l'Africa merita con urgenza un rifinanziamento sostanziale il negoziato quadro finanziario pluriennale deve identificare strumenti e meccanismi stabili ed efficaci di non minore portata rispetto a quello dedicato nel 2016 alla rotta del Mediterraneo orientale. Ciò significa, infatti, un approccio davvero integrato alle rotte del Mediterraneo. La riduzione degli sbarchi nel Mediterraneo centrale è, infatti, un risultato da preservare, ma non da sopravvalutare; vanno, infatti, tenute bene a mente sia la dinamica dei vasi comunicanti - che ora vede prevalere la rotta del Mediterraneo occidentale, ma domani chissà sia la fragilità della situazione libica o i complessi aspetti dei Paesi limitrofi, che possono riportare da un momento all'altro ad aumenti del flusso migratorio. Il caso libico è singolare, peraltro, perché propone all'Unione europea attori e interlocutori differenti rispetto ai protagonisti delle rotte del Mediterraneo orientale oppure occidentale. Tale aspetto rende ancora più necessario un approccio integrato ed equilibrato, anche in ordine al finanziamento e alla gestione della migrazione. Desidero soffermarmi sul Mediterraneo centrale anche per un altro aspetto cruciale del dibattito europeo sulla migrazione: l'aggiornamento del mandato dell'operazione Sophia, che l'Italia richiede fin dall'estate, per evitare che gli sbarchi dei migranti, salvati dalle navi dell'operazione, avvengano soltanto in Italia. Anche su questo tema occorre che tutti gli Stati membri si chiedano davvero se valga la pena di mettere in pericolo un'operazione di forte valenza politica, in primo luogo per la sicurezza del Mediterraneo, per reiterare una chiusura netta a un aggiornamento del mandato che l'Italia chiede allo scopo di ottenere finalmente uno sforzo condiviso sugli sbarchi. È prevista al Consiglio europeo una sessione su sicurezza e difesa in cui esaminare i positivi avanzamenti dell'Unione europea in tale settore, incluse le missioni di politica di sicurezza e difesa comune. Ebbene, una simile discussione va collegata a un impulso del Consiglio europeo affinché la questione dell'aggiornamento del mandato dell'operazione Sophia possa essere risolta in modo positivo e tempestivo. Per quanto concerne il quadro finanziario pluriennale, è prevista dal Consiglio europeo una discussione sul possibile obiettivo temporale per concludere un accordo che tradizionalmente richiede molto tempo e molta pazienza politica, oltre che tecnica. L'Italia ritiene che la tempistica non debba andare a scapito della qualità del negoziato. Dico questo perché, di fronte alle sfide che l'Europa ha davanti e riguardano da vicino la fiducia stessa dei cittadini nei confronti delle istituzioni europee, non possiamo prendere scorciatoie che conducano a un bilancio settennale - questa, come sapete, è la sua durata - inadeguato alla posta in gioco. L'Europa ha, infatti, bisogno di spendere meglio sia per le nuove priorità come migrazione, sicurezza, investimenti, ricerca che per le politiche tradizionali come la coesione e la politica agricola comune. Deve, inoltre, aprirsi alle nuove risorse proprie. I cittadini europei del prossimo decennio necessitano di un'Europa che abbia un effettivo valore aggiunto quando spende denaro del contribuente europeo. Questa esigenza, ormai ineludibile, riguarda sia le citate nuove priorità che strumenti come coesione e politica agricola comune, che garantiscono effettiva convergenza socio economica e sostegno agli imprenditori in un settore nevralgico, soprattutto per l'Italia e per le nostre economie esposte ad alcuni effetti della globalizzazione. Anche sul quadro finanziario pluriennale intendo riaffermare queste priorità italiane con l'orgoglio di un Paese che è il quinto contributore netto e che, da membro fondatore dell'Unione europea, reputa essenziale un negoziato all'altezza di un'Europa moderna. A questi temi si aggiungerà una discussione su temi non meno rilevanti, quali il completamento del mercato unico. Le conclusioni mirano a un segnale del Consiglio europeo a favore del completamento del mercato unico entro la fine dell'attuale legislatura. Da parte italiana si reputa essenziale che questo impulso vada anche in direzione del sostegno che l'Europa deve dare alle piccole e medie imprese. Quello della disinformazione è un tema complesso, su cui la discussione mira per il momento a dare una base di sostegno politico all'attività che la Commissione avvierà con un ambizioso piano d'azione congiunto appena presentato dalla Commissione stessa. Siamo, dunque, alle battute iniziali di uno sforzo europeo coordinato, che riteniamo necessario proprio in virtù della natura complessa e plurale del problema. L'Italia intende farsi portatrice di una visione secondo cui la sfida legata alle azioni di disinformazione, venendo da una molteplicità di soggetti, statuali e non, richiede un approccio strategico, multidimensionale e di ampio respiro che dia rilievo anche ai processi educativi e formativi per rafforzare la resilienza delle nostre società al fenomeno e non trascuri naturalmente i delicati profili di necessaria garanzia della libertà di informazione, fondamento essenziale delle nostre democrazie. Infine, mi soffermo sulle relazioni esterne. Su questo fronte l'agenda del Consiglio prevede la periodica informativa della cancelliera Merkel e del presidente Macron sullo stato di attuazione delle intese di Minsk in vista della decisione, a gennaio, sul rinnovo semestrale delle sanzioni settoriali nei confronti della Russia. L'Italia intende essere coerente con il proprio approccio rispettoso della questione europea, ma al tempo stesso convinto che le sanzioni non siano un fine in sé bensì uno strumento finalizzato ad avviare la soluzione della crisi Ucraina. A questo proposito, resta per noi prioritario, in questa fase di crescente tensione tra Mosca e Kiev, acuita nei giorni scorsi dagli attriti del Mar d'Azov, lavorare insieme ai nostri *partner* europei per favorire una distensione e riportare il confronto al tavolo dei negoziati. Nella parte dedicata alle relazioni esterne le conclusioni del Consiglio prenderanno anche atto dello scambio di opinioni dei *leader* quanto alla preparazione del *summit* tra l'Unione europea e la Lega araba, previsto per il 24 e il 25 febbraio 2019, che rappresenta di per sé un importante segnale politico di un'Europa chiamata ad affermarsi quale attore credibile e responsabile nell'ambito dello scacchiere internazionale. Per tale ragione e per le grandi sensibilità in gioco, ove gli aspetti della sicurezza, dello sviluppo e della gestione dei fenomeni migratori non sono avulsi dal contesto geostrategico, sarà importante porre particolare attenzione ai temi dell'incontro e ai possibili risultati, garantendo il giusto equilibrio tra ambizioni e seguiti. L'Italia intende proporsi come interlocutore privilegiato, data anche la sua vicinanza geografica per affrontare congiuntamente le sfide trasversali che percorrono il Mediterraneo allargato. Il tema del dialogo e della consultazione dei cittadini è un tema importante e non possiamo affrontarlo con un approccio meramente burocratico. Per questa ragione, il Governo italiano ha voluto esaminare approfonditamente le modalità con cui poter svolgere in modo efficace il tema e ha optato per un approccio di più ampio respiro, orientando cioè la consultazione avviata in queste settimane alla sensibilizzazione degli studenti sull'Europa. Infine, vi è il tema del cambiamento climatico. È previsto un riferimento, nelle conclusioni, a una strategia di lungo periodo dell'Unione sul cambiamento climatico da sviluppare nei prossimi mesi sulla base di una proposta della Commissione europea. Si tratta di un auspicio condivisibile che sta all'Europa tradurre in politiche concrete e sostenibili. La nostra linea su questo tema è molto chiara, anche dalla lettura del nostro contratto di Governo: noi siamo per la piena realizzazione dei contenuti dell'Accordo di Parigi. Permettetemi, adesso, a margine delle comunicazioni sul prossimo Consiglio europeo, di condividere con il Parlamento alcune considerazioni in vista di un altro passaggio importante nel confronto con le istituzioni dell'Unione europea. Domani mi recherò a Bruxelles per incontrare nuovamente il presidente Juncker e altri componenti della Commissione. L'interlocuzione con l'Unione europea, in questa fase così significativa per la vita politica, economica e sociale del nostro Paese, è fondamentale. In queste settimane non ho mai interrotto i canali del dialogo; ho lavorato per avvicinare le posizioni e per spiegare in tutte le sedi la coerenza della nostra manovra economica e i suoi effetti virtuosi nel medio periodo sul tessuto non solo economico, ma anche sociale. Non intendo certamente distogliere l'attenzione sui saldi finali di bilancio che - com'è noto - determineranno uno scostamento dal disavanzo primario. Ho anzi lavorato e sto continuando a lavorare, anche in queste ore che precedono il mio viaggio a Bruxelles, affinché siano puntualmente quantificati, con apposite relazioni tecniche, i costi delle misure, soprattutto di quelle a più rilevante impatto sociale e che maggiormente destano la preoccupazione dei nostri interlocutori di Bruxelles. Ho già più volte ricordato che nella legge di bilancio, attualmente all'esame qui al Senato, si interverrà, soprattutto a seguito delle modifiche che saranno apportate durante l'*iter* parlamentare, sulla spesa per investimenti, di cui peraltro presenterò domani un programma dettagliato. inoltre illustrato alla Commissione le riforme che il Governo ha realizzato e quelle avviate. Non andrò a Bruxelles con un libro dei sogni, ma presenterò uno spettro completo del progetto riformatore di questo Governo e, con il supporto di un approfondito lavoro istruttorio che ho personalmente e direttamente coordinato, mi confronterò sui numeri, nella consapevolezza di essere in possesso dei dati macroeconomici per dimostrare che la manovra economica del Governo è stata concepita conoscendo bene la realtà economica italiana ed è stata strutturata nei suoi contenuti per rispondere alle specifiche esigenze del Paese *(Applausi all'interno del perimetro tracciato dalle regole e dai vincoli di finanza pubblica che derivano dall'adesione all'Unione europea e dall'appartenenza al sistema dell'euro. Ma né domani a Bruxelles, né ancora di più oggi davanti al Parlamento, mi posso limitare a concentrare l'attenzione solo su meri dati contabili. Con le elezioni del 4 marzo, gli italiani hanno espresso una richiesta - direi un'urgenza - per arrestare l'impoverimento e e l'emarginazione causati dal lungo ciclo avverso della crisi economica e da un processo di globalizzazione che ha visto penalizzate ampie fasce della popolazione. Abbiamo assistito a una progressiva esclusione dai benefici della vita associata di un numero sempre più consistente di cittadini, fenomeno che ha rimesso in discussione diritti sociali che sembravano appartenere per sempre al patrimonio giuridico-sociale del nostro sistema democratico. Con il programma di Governo abbiamo quindi individuato responsabilmente le misure concrete per invertire con decisione questa tendenza. Il programma, accanto alle misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori, propone interventi di equità sociale necessari e anche sostenibili. È una risposta urgente ai diversi e molteplici bisogni primari dei cittadini. E se siamo stati costretti a procedere a uno scostamento dal *deficit* inizialmente previsto, lo abbiamo fatto non certo a cuor leggero, ma proprio per realizzare gli obiettivi che gli italiani chiedono con prepotente urgenza. Mi riferisco alle misure di equità sociale, di *welfare,* di sostegno al reddito, di semplificazione e pacificazione fiscale, di inclusione soprattutto in favore delle giovani generazioni, le quali hanno più pesantemente sofferto gli anni della crisi, perché sono state escluse dal mercato del lavoro, con conseguenze non solo economiche, ma tali da compromettere gravemente la qualità della loro esistenza. Questa è una manovra che farà crescere l'Italia, e non solo con riferimento al PIL, ma con riferimento al PIL integrato dal L'abbiamo costruita pensando allo sviluppo, alla crescita economica, alla modernizzazione delle imprese, all'innovazione tecnologica. Siamo convinti che tutto questo debba essere realizzato in modo sostenibile, conservando inalterato, per quanto possibile, l'ordito dei diritti sociali (dall'istruzione alla salute) ricevuto come preziosa eredità dalle generazioni che ci hanno preceduto. Certamente i diritti costano - come insegna Cass Sunstein - ma sono costi che le società democratiche devono sostenere se veramente credono nel primato della persona umana come valore che trascende e supera ogni altro interesse e che non può essere sacrificato per perseguire altri, pur legittimi, obiettivi. L'Italia è stata protagonista nei passaggi decisivi della storia dell'integrazione europea, ha sempre partecipato in senso inclusivo e solidale alla soluzione delle crisi politiche ed economiche che hanno vissuto gli altri Stati membri. Crediamo e siamo parte integrante dell'Unione europea. Per questa ragione stiamo cercando di compiere tutti gli sforzi per diradare le perplessità sollevate dalla Commissione. Ci siamo adoperati per illustrare puntualmente i nostri obiettivi, rivendicando il diritto di effettuare una manovra di carattere espansivo, con interventi di spesa e investimenti programmati per stimolare la crescita e la produttività e per garantire la stabilità non solo finanziaria, ma anche sociale. Siamo nel mezzo di un confronto serrato, che confidiamo essere leale e paritario, nell'auspicio che - come sempre accade nelle trattative - si possa trovare un punto di equilibrio e di convergenza. Resto fiducioso nel buon esito del dialogo.

Signor Presidente, la tirannia dei tempi, che è comprensibile vista l'organizzazione dei nostri lavori, ci impone di fare riflessioni

Basta vedere ciò che capita in Francia per capire che in Europa stiamo vivendo tempi particolarmente difficili.

dal 49 al 64 per cento. Mi auguro - sono convinto - che questa maggioranza voglia tenere nella massima considerazione questo *sentiment* collettivo. sono preoccupato per l'epilogo che rischia di avere la vicenda della Brexit, che dimostra come sia stata assai avventata la scelta fatta nel Regno Unito. Unito. Signor Presidente, io mi auguro che nella trattativa sulla Brexit, che è il primo punto che lei ha riferito, ci sia la necessaria severità, unita alla flessibilità, perché il Regno Unito è e rimarrà storicamente uno

Resta un piccolo particolare: mi auguro che sulla redistribuzione la sua battaglia abbia la meglio sulla resistenza dei Paesi che parte di questa maggioranza ha scelto come Paesi amici a livello europeo. se prevalessero le tesi dei Paesi del Gruppo di Visegrád, noi non faremmo alcuna redistribuzione. Lei, giustamente, nel richiedere il rigoroso rispetto di alcuni principi, ha praticamente delineato una piattaforma alternativa a quella di alcuni Paesi. Io sto con lei, non sto con quei Paesi. Sono un patriota e un italiano e voglio che prevalgano le sue opinioni.

riguardante la Russia. Voglio dire solo una cosa. Chiedo alla maggioranza di evitare di parlare contro le sanzioni salvo poi, alla fine, doverle sottoscriverle. lei ha ragione: le sanzioni sono non un fine, ma uno strumento. Cerchiamo di avere equilibrio, perché non credo che nemmeno i nostri *partner* russi possano condividere molto l'atteggiamento di chi cambia orientamento dal mattino alla sera, dicendo di essere contro, salvo poi

Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione «Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile». Nei giorni scorsi il ministro Salvini - lo capisco, perché i comizi li abbiamo fatti tutti e, quindi, non voglio non voglio innescare una polemica su una frase, appunto, da comizi - ha detto che vuole trattare con l'Europa in rappresentanza di 60 milioni di italiani. a trattare con l'Europa ci va il Presidente del Consiglio. Questo Presidente del Consiglio ha tenuto aperto il canale di dialogo. Oggi siamo alla fine del film.

vada Bruxelles non solo per illustrare i contenuti della manovra, che è nel suo diritto-dovere di farlo, e non solo per tenere i canali di dialogo aperti, ma anche per evitare in ogni modo una procedura di infrazione che renderebbe vulnerabile all'aggressione dei mercati il nostro Paese, che deve collocare i titoli del debito pubblico sul mercato. Penso quindi che in questo momento

tutte le polemiche sbracate contro Juncker, contro questo e quell'altro? Servono a fare una propaganda permanente che nuoce all'Italia sui mercati internazionali. Chiedo e credo

le auguro successo in entrambe le sue missioni a Bruxelles: quella di partecipazione al Consiglio europeo e quella di negoziato con la Commissione europea. Le sue comunicazioni sono state, come sempre, molto chiare; chiare le comunicazioni, ma tutt'altro che chiara è la politica del suo Governo, in particolare sui due temi da lei toccati oggi: la manovra economica e la politica europea dell'Italia. Quando il ministro Tria, il 28 novembre, ha illustrato in quest'Aula gli elementi di novità previsti per la manovra rispetto alla precedente impostazione del Governo, ho dichiarato di considerarli non già come segni di cedimento alle osservazioni dell'Unione europea o alle pressioni dei mercati, ma al contrario come segno di un'evoluzione verso una strategia più matura, sia pure su una manovra per la quale il mio giudizio complessivo resta negativo, perché non gioverà né all'occupazione né al risanamento della finanza pubblica. Mentre però lei fa un lavoro che - come il presidente Casini ha appena sottolineato - va nell'interesse dell'Italia, c'è una sorta di «schema Penelope» per cui altri distruggono quotidianamente - non so se di giorno o di notte, nel caso di specie - il lavoro che fa. Si è trattato di gravi errori di posizionamento dell'Italia in Europa e di gravi errori nel modo di rapportarsi con essa. Ho definito un passo avanti e non indietro dal punto di vista economico la revisione della manovra. Ma non nascondiamoci che dal punto di vista della politica europea dell'Italia, l'insieme del primo e del secondo tempo sono stati una Caporetto politica: nel primo tempo i due Vice Presidenti del Consiglio hanno fatto a gara con affermazioni «Me ne frego dell'Europa, non ci muoveremo di un millimetro», «Se Bruxelles ci boccerà, vuol dire che stiamo facendo le cose giuste» e via di seguito. E poi un docile secondo tempo: «Il Governo è pronto a modificare la manovra, l'importante è evitare la procedura di infrazione». Lei ha esperienza ormai e conosce la storia; sono esattamente questi voltafaccia che, nel corso dei decenni lontani e dei secoli, hanno costruito nella visione delle potenze straniere l'immagine di un'Italietta che abbaia, ma non morde. Bisogna non abbaiare,

solo il gusto di non prendere seriamente le sue minacce e qualche volta il piacere di metterla sotto. Alla luce di tutto questo, ci manca solo che l'Italia dia a un Vice Presidente del Consiglio, che in un eccesso di entusiasmo l'ha invocato, il mandato per trattare con l'Europa. La mia ultima considerazione è che lei però, signor Presidente del Consiglio - come ha ricordato di nuovo il senatore Casini - ha gli strumenti, perché la Costituzione le dà il modo - ma io mi permetto di dire anche che le impone - con l'articolo 95, di dirigere la politica generale del Governo, della quale lei è responsabile. I Ministri, fossero anche Vice Presidenti del Consiglio - come dice la Costituzione - sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro Dicasteri. Se - per esempio - un Ministro dell'interno, con proprie dichiarazioni, plasma la politica estera dell'Italia, così come viene percepita poi dalla stampa internazionale e ripercossa nelle altre capitali, non solo un *vulnus* - che io non so come lei faccia a tollerare - al Presidente del Consiglio, al Ministro degli affari esteri e qualche volta al Ministro per gli affari europei, ma anche un *contempt of parliament*, perché le due Camere vengono di fatto espropriate della possibilità di di concorrere a formulare e a sorvegliare la politica estera del Governo. Faccio parte della Commissione affari esteri del Senato, dove sentiamo di tanto in tanto le diligenti esposizioni del Ministro degli affari esteri; ma è chiaro che non è lui a fare la politica estera dell'Italia. Quindi io credo che, per una questione di funzionalità, occorra proprio evitare all'Italia andamenti così oscillanti da distruggere quello che viene costruito e, anche per rispetto del Parlamento, facendosi forza, lei si avvalga più pienamente del diritto, ma anche del dovere, che la Costituzione le dà di dirigere la politica generale del Governo. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, presidente Conte, il prossimo vertice del Consiglio europeo, ormai alle porte, è un'importante occasione per far soffiare, anche in Europa, il vento del cambiamento. La maggioranza politica che sostiene il Governo è compatta e vuole davvero un'Europa che possa avvicinarsi alle reali esigenze dei cittadini e essere al servizio del bene comune dei suoi cittadini. Non chiediamo grandi cose, signor Presidente, ma il cambiamento è prima di tutto un nuovo modo di pensare alla politica: è invertire le priorità, per mettere al centro il cittadino. Questo può esporci a critiche, ovviamente, ma non ci fermeremo mai. Per me cambiamento in Europa significa dare più importanza al bilancio sociale che a quello finanziario e prendere atto che è ora di fare politiche che promuovano la crescita economica. Dobbiamo essere realisti, signor Presidente: l'*austerity* in Italia non ha diminuito il debito pubblico e ha messo in secondo piano la lotta alla povertà che è un obiettivo perseguito dalla stessa Unione europea. In questo intervento mi limiterò a esporre al Presidente del Consiglio alcuni punti che ritengo fondamentali per un vero cambiamento in Europa, soprattutto per il nostro Paese. Per quanto riguarda l'ambito economico e lavorativo, anzitutto occorre evitare che aumenti ulteriormente la pressione fiscale sui contribuenti nazionali. Aumentare l'IVA può compromettere l'efficacia delle nostre riforme, perché l'aumento di tasse rallenta i consumi e la crescita. Questo lo dice la legge dell'economia. Occorre poi impegnarsi nel contrasto alla povertà: è indispensabile che i fondi europei prevedano risorse per ostacolare la povertà perché, se l'obiettivo è il bene comune, non possiamo dimenticarci degli ultimi. Occorre poi rafforzare il programma COSMEriservato al sostegno delle piccole e medie imprese e facilitare l'accesso al credito. Non dimentichiamo mai il grande sforzo e gli immensi sacrifici delle nostre piccole e medie imprese nel difficile periodo della crisi economica. Abbiamo il dovere di credere che il loro sviluppo sia fondamentale per la crescita economica del Paese. Signor Presidente, la revisione dei parametri per la concessione di finanziamenti alle piccole medie imprese. L'Europa, quindi, deve proporre una revisione degli accordi di Basilea che non ostacoli la crescita attraverso l'agevolazione delle piccole e medie imprese, spina dorsale del nostro Paese**.** Non dimentichiamo, infine, i giovani: la disoccupazione giovanile è molto elevata, è un indice di una società malata. Dal futuro dei giovani dipende il futuro dell'Europa e, in particolare, del nostro Paese, che ha sofferto di più: occorre potenziare le politiche attive del lavoro e la formazione professionale per consentire un consentire un collegamento strategico tra scuola e imprese. Anche questa è una scommessa importante per l'Europa. Sul tema del mercato unico, signor Presidente, occorre un impegno comune perché questo mercato porti benefici ai cittadini e alle imprese, e non una riduzione delle possibilità lavorative o delle tutele sociali. La concorrenza sana è quella che non solo guarda al costo del prodotto, ma che tutela anche e soprattutto i diritti dei lavoratori: il mercato unico non deve trasformarsi in una corsa al ribasso, ma deve promuovere le efficienze e rimuovere le inefficienze a vantaggio dei cittadini e delle imprese. Occorre guardare al mercato unico nella consapevolezza del nostro tessuto socio-economico, fatto di piccole e medie imprese di qualità che danno lavoro a milioni di cittadini italiani. Proprio per questo è importante sostenere il rinnovamento dei loro processi produttivi ed evitare che restino schiacciate dai colossi del mercato. Altro punto chiave è la lotta alla delocalizzazione fiscale: il principio di libera circolazione delle imprese non deve condannare alla precarietà i lavoratori. Ogni impresa è fonte di vita per le famiglie e, nel mercato comunitario, non si può consentire che la delocalizzazione avvenga per aumentare i profitti risparmiando sul costo del lavoro. Il costo del lavoro è composto dai diritti: e se ci sono Paesi in cui i diritti sul lavoro mancano, è lì che bisogna intervenire perché il mercato migliori e perché la concorrenza sia sana. L'Europa ha fortemente bisogno di coesione: il mercato unico deve essere rafforzato per affrontare l'inevitabile sfida futura e imminente proveniente dall'Est del mondo, e deve essere un modello competitivo fondato sui diritti e sul rispetto della dignità umana. Sul tema dell'immigrazione, il contrasto alla tratta degli esseri umani necessita di un intervento comunitario, mediante direttiva o regolamento, che consenta una strategia comune per fermare sia gli scafisti che tutti coloro che hanno fatto dell'immigrazione un *business* sulla pelle di tanti esseri umani. umani. È necessario promuovere e rafforzare i rapporti con le istituzioni africane e potenziare lo scambio di informazioni tra l'Europa e l'Africa.

Promuovere lo sviluppo dell'Africa è un investimento per il mondo intero. Signor presidente Conte, concludo il mio intervento incoraggiando il Governo del cambiamento a continuare su questa strada e a restare sempre dalla parte dei cittadini. È per questo che siamo stati eletti ed è per questo che siamo qua. È un percorso importante verso il rinnovamento di un'Europa che sia vicina al popolo, che faccia il suo interesse e lavori per la sua sicurezza. Questa è l'Europa che vogliamo. Questo è il futuro dei cittadini europei

*(Misto-LeU)*. Signor Presidente del Consiglio, il Consiglio europeo che si riunisce a Bruxelles domani e giovedì non è soltanto il terzo a cui lei partecipa, ma cade in un momento di grandissima difficoltà per l'Unione Ancora più dei casi specifici, come la Brexit, la situazione in Francia o anche il contenzioso con il nostro Paese, questa situazione di *impasse* è ormai segnalata chiaramente dall'impossibilità di procedere sulla strada del bilancio comune europeo e di un'unione bancaria fondata sulla condivisione

nel 2018. Questi sono i risultati dell'impossibilità di trovare soluzioni comuni. Tutto ciò è conseguenza diretta del prevalere degli egoismi nazionali e degli interessi parziali sull'interesse comune dell'Unione europea. A questa prevalenza ottusa degli egoismi nazionali e nazionalisti il nostro Governo - anzi, il suo Governo - ha contribuito e continua a contribuire. Non è un caso che, oggi, i Paesi che più insistono per punire la violazione delle regole del rigore da parte dell'Italia sono proprio quelli politicamente più vicini al Governo italiano, ovvero i Paesi dichiaratamente sovranisti, che dicono «prima gli austriaci», «prima gli ungheresi» e così continuando. Per questa strada, imboccata anche dal suo Governo, l'Unione europea non correggerà i propri enormi limiti, che sono la causa principale della situazione di difficoltà e anche di sofferenza nei vari Paesi, e che rischia di portare ancora una volta alle estreme conseguenze. Gli stessi errori e la stessa strategia controproducente hanno determinato, nella discussione sulla legge di bilancio, una situazione assurda e inaudita.

di bilancio e quali sono e come sono progettate nei particolari essenziali le misure cardine. Tra l'Italia e l'Unione europea è in corso quindi una trattativa, il cui esito potrebbe avere però delle conseguenze di straordinario impatto sulla vita degli italiani. Il suo incontro di domani con Juncker dovrebbe quindi essere uno snodo decisivo. I tempi sono ormai esauriti, ma dei contenuti della trattativa, arrivata ormai alla fase finale, il Parlamento non è al corrente, ne è tenuto all'oscuro. Anche oggi, signor Presidente, nella sua comunicazione si è limitato ancora una volta a fornire *slogan* buoni per tutti gli usi. Trincerandosi dietro un'estrema vaghezza, non ci ha detto nulla su quale sarebbe l'oggetto del confronto serrato di cui ha parlato. Non ha indicato neppure per sommi capi quale sia quel punto di equilibrio e convergenza che lei si augura - non si capisce bene con quanto fondamento - di poter raggiungere. Questa situazione che è paradossale e anche pericolosa - ve ne rendete perfettamente conto - purtroppo è il risultato di una strategia fallimentare che avete adottato nei rapporti con l'Unione europea. Non intendo dire - e lei lo sa perfettamente - che avreste dovuto accettare supinamente le regole rigoriste; anzi, al contrario, nessuno più di noi ha criticato la miopia e la pericolosità dell'*austerity*, che ha reso intollerabili le condizioni di vita di milioni di cittadini in Italia e in Europa. Il problema avrebbe dovuto essere posto,

avrebbe potuto e dovuto trovare alleati. Avrebbe dovuto e potuto dar vita a un fronte in grado di incidere davvero in profondità sulla struttura e sugli errori dell'Unione europea. Invece l'Italia, signor Presidente, in questo momento si trova isolata come mai era successo in precedenza, e quindi è più debole di quanto non sia mai stata. L'Italia avrebbe dovuto e potuto sforare il *deficit* concordato, ma mettendo in campo un progetto credibile di sviluppo basato su investimenti mirati da contrapporre alla cecità del rigorismo di Maastricht e del *fiscal compact*. Ha preferito invece puntare sulla propaganda, su una manovra fintamente espansiva che rispondeva esclusivamente alle esigenze della propaganda a breve in vista delle elezioni europee. Allo stesso modo, ha adottato toni bellicosi, provocatori, sempre sull'onda della propaganda - come negli ultimi giorni e ore - del suo Vice *Premier*, dei quali oggi però noi continuiamo a pagare il prezzo nelle trattative con l'Europa, alle quali, dopo tanto aver ruggito, il Governo - ne ho paura - dovrà adeguarsi, ma al ribasso, signor Presidente, oggi molto più di come poteva essere un mese fa. Voi avete messo l'Italia in una situazione estremamente rischiosa su molti piani: dalla minaccia di una procedura d'infrazione molto pesante a quella di un collasso anche molto forte sul fronte bancario. Non è un mistero per nessuno che proprio la vostra politica sia uno degli alibi messi in campo per bloccare quei passaggi fondamentali di cui parlavo prima. È ora, però, che vi decidiate a uscire dalla propaganda e a rivedere le posizioni, e non per adeguarvi alle regole dell'austerità, ma per modificarle davvero; in caso contrario, riuscirete non solo a smantellare la stabilità finanziaria, ma anche

sobrietà. Fratelli d'Italia, che il Tricolore ha da sempre nel proprio DNA, in questi momenti è con il Governo, è vicino al Governo. Ci auguriamo però che lei possa andare a quell'incontro con la schiena dritta. Non vorremmo si ripetessero le schiere di Governi della sinistra,

Io non condivido - e con me il Gruppo Fratelli d'Italia - gran parte della manovra economica, della quale lei, Presidente, dovrà discutere in sede europea; ma, pur non condividendola, mi auguro che lei sappia esserne interprete con fierezza, a dimostrazione che

che questa posizione non sia, poi, così chiara e coerente. Temo che, guardando alla politica estera come alla politica interna, il Governo cosiddetto del cambiamento non abbia davvero il coraggio di essere il Governo del cambiamento. Mi è dispiaciuto che, su un tema come il Global compact, si siano sentite voci differenti, dissonanti, e che un Governo che vuole porre un limite un limite al fenomeno migratorio, che gravi ripercussioni ha avuto non solo sul piano sociale, ma anche sul piano economico, non abbia espresso con fermezza una posizione contraria ai principi insiti nel Global compact e non abbia, quindi, seguito quella strada che gli Stati Uniti o l'Australia e finanche i Paesi di Viségrad hanno, invece, chiaramente enunciato. Mi sarei aspettato dall'Italia, da questo Governo del cambiamento, una posizione più chiara su questo argomento. Venendo agli aspetti economici, il tempo è poco e mi limito a qualche assunto.

quando tutte le categorie economiche, dalle piccole alle grandi, per arrivare ai professionisti, esprimono negatività su questo percorso, allora l'indebitamento del quale l'Europa ci incolpa può davvero diventare una colpa.

Grazie a tutti di sviluppo, di cambiamento, e mai sia supina alle posizioni di quei tecnocrati che a Bruxelles hanno malamente governato l'Europa e malamente influito, grazie a chi ci ha preceduto, sulla politica economica dei Governi precedenti.

alla partenza per una missione di particolare importanza. Ricordo che, oltre che rappresentante del secondo Paese manifatturiero in Europa, nonché uno dei membri fondatori dell'Unione europea, è anche rappresentante del Paese che ha più cittadini sparsi in Europa. Mi riferisco, in particolare, a oltre 3 milioni di cittadini italiani che risiedono regolarmente in Europa: non c'è nessun altro Paese dell'Unione europea che ha queste caratteristiche. pertanto, avrà una responsabilità particolare anche nei confronti di questi nostri cittadini residenti in Europa. Molti di questi risiedono nel Regno Unito: oltre 700.000, dai dati delle autorità inglesi, mentre è un dato molto sottostimato quello delle autorità italiane (380.000). Per coloro che risiedono in Inghilterra, l'ipotesi del *no deal*, dell'uscita dall'Unione europea del Regno Unito senza accordo, è una vera e propria sciagura. Al riguardo, la inviterei a segnalare alle autorità del Governo inglese l'opportunità di procedere a un secondo *referendum*, per uscire dall'*impasse* in cui si sono messi.

è pronto per essere considerato). Quindi, dovrà esporre alle autorità europee la compatibilità tra i vincoli politici che derivano al Governo dal contratto di programma (che sono ben chiari a tutti), a tutti), i vincoli che ci derivano dall'appartenenza all'Unione europea - che noi abbiamo iscritto nella Carta costituzionale - nonché i vincoli debitori che ci derivano dalla nostra posizione peculiare sui mercati internazionali. Già riuscire a trasmettere questo messaggio di presa di coscienza tardiva, ma piena del Governo italiano che lei rappresenta della compatibilità tra questi tre tipi di vincoli diversi sarebbe un passo avanti molto benvenuto. La garanzia dell'ordito dei diritti sociali - che lei con bella espressione ha ricordato - deriva dalla compatibilità di tutti e tre questi vincoli. Nello specifico, il Consiglio europeo si occuperà di una serie di questioni tecniche e, soprattutto, del quadro finanziario pluriennale (QFP). A riguardo, viene richiesto ai Paesi europei, anche a causa del recesso - se ci sarà del Regno Unito, di aumentare le risorse a disposizione. Lei ha citato l'Italia come quinto contributore netto. Credo che, in realtà, noi siamo già il terzo. Una volta uscito il Regno Unito, saremo il terzo contributore netto. Siamo rimasti solo in tre Paesi all'interno dei 27 a dare di più di quanto ricevono. Questo sarebbe il caso di ricordarlo alle autorità e agli eurocrati di Bruxelles. Germania e Francia, che sono gli altri due Paesi che hanno questa caratteristica, hanno ritorni di vario tipo, che noi sembra non riusciamo a ottenere. In coerenza con la Strategia europea 2020 cambieranno le rubriche e le ripartizioni tra programmi. Noi condividiamo con la Commissione europea l'aumento dei fondi per la ricerca, l'innovazione e l'agenda digitale (115 miliardi) e quelli per i giovani. È previsto il raddoppio dei fondi Erasmus a 30 miliardi. Ricordo che Erasmus è stata citata da un sondaggio dei cittadini dell'Unione europea, insieme alla UEFA Champions League e alle linee aeree *low cost*, come i tre fattori determinanti che hanno fatto crescere l'Europa e la sensazione di appartenere all'Unione europea tra i cittadini.

tedesco, ma sembra che non siamo stati in grado di fare breccia: 35 miliardi, di cui 10 per il fondo asilo e migrazione e circa 22 per la gestione integrata delle frontiere, sono veramente troppo pochi. Basterebbe paragonarli ai circa 90 per la cooperazione internazionale. C'è - mi sembra - una scarsa cognizione a livello europeo dell'importanza che una gestione porosa e diversificata delle frontiere esterne causa all'Unione europea. Non mi riferisco tanto e solo alle migrazioni umane, quanto al traffico delle merci. Presidente, una volta che le scarpe o i prodotti agroalimentari illegali dell'estremo Oriente entrano da un porto olandese, tedesco e greco e poi circolano liberamente all'interno del mercato europeo sono i nostri produttori di *made in Italy* di qualità a patirne le conseguenze. Le frontiere comuni devono essere un problema comune finanziato e gestito in maniera comune, effettiva e uniforme. Non c'è tempo per parlare di altre cose, ma ci tengo a terminare con un accenno alla politica sulla condivisione dei rischi, che lei ha citato. La proposta di regolamento relativa a un sistema europeo di assicurazione dei depositi depositi per l'istituzione di un Fondo monetario europeo, in base alla quale il Fondo monetario europeo potrebbe costituire il meccanismo di *backstop* (garanzia) comune per il fondo di risoluzione unico delle crisi bancarie e fungere da prestatore di ultima istanza al fine di facilitare la risoluzione ordinata delle banche in difficoltà senza ricorrere al denaro dei contribuenti, a differenza di quanto è stato fatto in passato, è in realtà un'antica proposta di Forza Italia del ministro Tremonti. Noi siamo contenti. Ci fa piacere che il tempo e i *partner* nordeuropei ci diano finalmente ragione a riguardo. *(Applausi

Signor Presidente, presidente Conte, signori del Governo, colleghi, il Consiglio europeo dei prossimi giorni è un appuntamento a cui dobbiamo presentarci preparati, in vista di un rassicurante futuro non solo per l'Italia ma soprattutto per l'Unione europea. Non è facile confrontarsi su temi quali quelli da lei illustrati; temi di scottante attualità, di indiscusso interesse, ma su cui potrebbero verificarsi incomprensioni tali da non consentire un vero e proficuo dialogo tra le parti. Allora, la nostra voce in Europa deve essere forte, ma in particolare deve essere chiara su quanto andiamo a discutere e su cui è evidente che dobbiamo mediare. In un precedente incontro, lei, presidente Conte, parlando del bilancio pluriennale, che contiene le indicazioni fondamentali del bilancio europeo per i prossimi anni, ha detto che l'Italia è un contribuente netto al bilancio dell'Unione per significare che l'Italia ha ottenuto assegnazioni di entità inferiore rispetto alle contribuzioni che versa al bilancio comunitario. Tutto questo è stato certificato dalla Corte dei conti nella relazione annuale al Parlamento sui rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei fondi comunitari, dove si precisa che quella di contributore netto è una posizione nella quale il Paese si trova da molti anni. Proprio in virtù di questo, dobbiamo insistere sulle potenzialità dell'Italia per una crescita positiva dell'Europa: sull'aumento delle risorse finanziarie nei settori della ricerca, dell'innovazione, della formazione formazione dei nostri giovani; della migrazione, della sicurezza interna e della difesa, dell'ambiente. Dobbiamo difendere meglio le politiche agricole e le politiche di coesione, non permettendo più tagli in alcuni dei settori fondamentali per l'economia del nostro Paese. In questa prospettiva dobbiamo pensare a un mercato unico più equo, allo sviluppo concreto del potenziale del mercato unico e a una sua maggiore integrazione per ottenere benefici per tutti i cittadini europei. Adottare la strategia del mercato unico significa migliorare la competitività dell'economia europea creando nuove opportunità per le imprese e i consumatori. Per questo dobbiamo lavorare in Europa: per rimuovere ogni ostacolo alla libera circolazione di beni e servizi; per espandere le possibilità di crescita economica e occupazionale, anche nel nostro Paese. pretendere il rispetto adeguato ed efficace delle norme esistenti per giungere a una sintonia tra le prescrizioni europee e quelle dei Paesi membri, con iniziative politiche mirate che, riconoscendo a ogni Nazione le proprie specificità relativamente ad alcuni settori economici prioritari, consentano il raggiungimento del benessere di tutti. Per le piccole e medie imprese, le politiche di contrasto alla delocalizzazione fiscale che vogliamo portare avanti sono, appunto, mirate e rafforzare la loro competitività in Europa, focalizzando gli investimenti verso una politica industriale innovativa, intelligente e sostenibile. Sempre in tema di mercato unico, bisogna condividere a livello europeo le misure di tassazione omogenea di ogni attività produttiva e non solo dell'attività digitale e dei servizi, priorità assoluta dell'Unione europea, con proposte normative valide e ricerca di soluzioni efficaci. Signor Presidente, comprendo che questo costituisca uno sforzo eccezionale, ma è uno sforzo necessario e condivisibile per evitare nuove distorsioni che devono essere conosciute e analizzate proprio affinché queste ultime non abbiano più rilievo di quanto si cerca di correggere. Altro importante tema è quello della migrazione, per cui è necessaria una cooperazione europea non solo per migliorare la normativa di regolamentazione dei flussi migratori, ma per incentivare e promuovere azioni risolute di contrasto alle reti criminali che sfruttano i migranti indifesi. Il traffico dei migranti è diventato una forma di criminalità sempre più violenta, con vere e proprie violazione di diritti umani. impegnarsi veramente per potenziare la cooperazione; condividere i dati in possesso degli Stati per ottimizzarli; incrementare i rapporti positivi con i Paesi di origine e di transito; condividere le informazioni e la cooperazione giudiziaria e di polizia sul traffico dei migranti; promuovere iniziative e progetti di sviluppo con l'obiettivo di contrastare il traffico di migranti, e infine insistere per la riforma del Regolamento di Dublino, che permette ancora di addossare allo Stato di prima accoglienza tutti gli oneri che riguardano i migranti; collaborare, invece, per rinnovare l'esistente, con un coinvolgimento attivo di tutti i Paesi europei. Sul fronte delle relazioni esterne, signor Presidente, è opportuno che il nostro Governo si impegni a lavorare sul piano europeo per gli investimenti esterni, promuovendo investimenti strategici anche a livello continentale e nazionale, soprattutto nel campo dell'istruzione e delle competenze, attraverso borse di studio e programmi di scambio, rinvigorendo il contesto imprenditoriale, intensificando il dialogo per una migliore integrazione economica e gli scambi commerciali, trovando spazi di confronto con la Federazione russa, per evitare l'inasprimento di relazioni internazionali fondamentali e garantire sempre la difesa dell'Europa, mantenendo stabile e forte la politica europea di vicinato, consolidando i concetti di democrazia, diritti umani, Stato di diritto, buon Governo e i principi di economia di mercato e sviluppo sostenibile. Signor Presidente del Consiglio, sicura che lei saprà ben rappresentare l'Italia in Europa, ricordi all'Europa che noi siamo uno dei Paesi fondatori e che nel progresso dell'Unione abbiamo posto la speranza di un futuro favorevole, non solo sotto l'aspetto socio-economico, ma anche e soprattutto di pace e collaborazione. Faccia comprendere ai nostri *partner* che l'Italia è Europa e, con questa consapevolezza e nella certezza che questo sia un sentimento comune, rappresenti le esigenze del popolo italiano con la moderazione che la contraddistingue, ma con la fermezza di chi sa che ha il pieno sostegno del Parlamento e dello Stato intero.

dirò più avanti sulla Brexit, ma vorrei preannunciare una posizione chiara: io penso che non si debba riaprire il negoziato, riaprire il negoziato, perché sarebbe un pericolo e un rischio enorme. Non ripetiamo lo stesso errore che fu fatto con Cameron. Sul bilancio pluriennale, direi che è persino scontato che l'Italia difenda i suoi interessi maggiori, cioè le risorse per i fondi strutturali e la politica agricola comune,

l'Unione europea a rispondere a tutte le sfide a cui è chiamata, avendo un bilancio di 160 miliardi di euro all'anno, che corrisponde all'1 per cento del reddito nazionale lordo e al costo di mezza tazza di caffè al giorno per ogni cittadino italiano.

di aumentare i fondi per l'innovazione e per la ricerca - cosa giustissima - e poi non voler provare a fare la cosa più giusta, cioè fare la riforma del bilancio comunitario. Io vi chiedo di sostenere sostenere le proposte che ci sono in campo. *(Applausi dal Gruppo PD)*. L'altro giorno una grande personalità come Piketty, insieme a tante altre personalità, ha offerto ulteriori proposte in questo senso, ma noi abbiamo la proposta del presidente Monti, sul tavolo europeo, ma che non viene esaminata adeguatamente. Lì c'è tutto. Abbiamo parlato, in questi anni, di *eurobond*, di *carbon tax*, di tassa sulle transazioni finanziarie, approvata dal Parlamento europeo, che giace in Consiglio. Presidente Conte, quando va a Bruxelles, può chiedere ai suoi colleghi perché la tassa sulle transazioni finanziarie, approvata dal Parlamento europeo, non viene attuata?

disponibili a farlo. Ognuno si assuma le proprie responsabilità. Questo dibattito sull'adeguatezza del bilancio si collega all'altra grande questione, che sarebbe un peccato se fosse rinviata a dopo le elezioni europee, cioè quella della *governance* economica e finanziaria della zona euro. Mi riferisco cioè alla possibilità di avere un bilancio comunitario con una capacità fiscale,

le grandi infrastrutture materiali e immateriali, l'innovazione, la ricerca, le grandi questioni sociali, ma anche l'innovazione legata a ciò che avverrà nei prossimi anni. Nel 2019 ognuno di noi avrà sei o sette aggeggi tecnologici; oggi ne abbiamo due o

necessarie a stare in un mercato del lavoro che sarà profondamente rivoluzionato da questa innovazione tecnologica. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Queste sono le grandi questioni che a livello europeo possono essere affrontate se ci sarà un bilancio adeguato e una nuova *governance* che preveda un Ministro del tesoro europeo e un Tesoro europeo con una capacità fiscale.

vogliamo ridurre l'immigrazione illegale, apriamo canali legali alla migrazione economica, altrimenti sono prese in giro per gli italiani. ultimo, torno sulla Brexit e sulla legge di bilancio. Sulla Brexit sono ore drammatiche: quello che sta succedendo nel Regno Unito dovrebbe essere di lezione per tutti e la parola «*exit*» dovrebbe essere espunta dai vocabolari, almeno da quelli europei. Ricordate sempre

versi e per certo tempo, ha sostenuto l'idea fallace della Italexit, della Brexit o della Grexit. Sul disegno di legge di bilancio, presidente Conte, lei ci deve portare un'intesa che consenta di scongiurare il rischio della procedura d'infrazione per l'Italia sul debito, che è cosa diversa e ben più grave della procedura sul *deficit*.

lei non deve rimanere con il cerino acceso perché il suo Governo è diviso e perché ci sono, da un lato, ammiccamenti e, dall'altro, polemiche nei confronti dell'Unione europea. Lei si deve assumere la sua responsabilità di Presidente del Consiglio ministri e portare a casa un risultato per il nostro Paese. Infine, guardiamoci intorno, colleghe e colleghi. La Francia è in ginocchio,

Non so se a voi questo mondo dà qualche piccolo, piccolissimo senso di preoccupazione e timore. A noi del Partito Democratico sì ed è anche per questo che vogliamo rafforzare coerentemente e concretamente, come ci ha insegnato e ci insegna il presidente Giorgio Napolitano, la nostra seconda patria: la patria europea.

potenziare, estendere e rendere più efficace ed efficiente la gestione dei fondi europei che sostengono le politiche di *welfare* degli Stati membri. non c'è solo l'aspetto economico. È un'Europa sempre meno matrigna e sempre più capace di sostenere la famiglia e le nuove generazioni, le uniche capaci

rafforzando i programmi e stanziando ulteriori somme per il COSME per programmare e parlare di piccola e media impresa, aiutando una cultura imprenditoriale a livello europeo.

i singoli Paesi, in quanto non siamo tutti uguali. Aumentando e valorizzando le differenze possiamo riuscire ad avere un'Unione europea grande e importante, altrimenti siamo tutti uguali. In tema di migrazione, penso che il nostro Paese abbia fatto veramente la sua parte. Infatti, ci sono non solo l'aiuto alle persone che arrivano qua, a cui dobbiamo dare una mano cercando

e parlare con una voce unica. Ci rendiamo conto però che queste sanzioni oggi danneggiano le piccole e medie aziende italiane. Per quanto riguarda l'Africa, la pacificazione e lo sviluppo del Corno d'Africa possono assicurare condizioni di vita migliori alle popolazioni locali, contribuendo alla stabilizzazione dei rapporti internazionali. Concludo dicendo - e su questo Presidente la stimo molto - che ogni tanto il no serve per far crescere. Come il babbo e la mamma dicono no per aiutare i figli, ogni tanto anche l'Italia deve dire qualche no per far crescere l'Unione europea. Quando è ora di dire sì, lo diciamo, e quando è ora di dire no, dobbiamo dirlo e avere il coraggio di farlo per la crescita.

*(FI-BP)*. Presidente Conte, tra due giorni lei si recherà a Bruxelles e incontrerà i Capi di Stato e di Governo dei Paesi europei, che viaggiano a velocità completamente differenti tra di loro. È di pochi giorni fa la pubblicazione da parte della Banca d'Italia che confronta le statistiche della finanza pubblica dell'Unione europea. Immagino che lei le abbia lette e notato quali differenze abissali vi sono tra i diversi Paesi dell'area Euro e dell'area

più di ogni analisi sociologica, la ragione della rivolta dei cosiddetti *gilet* gialli di questi giorni, ma anche la ragione della scelta dell'Irlanda quale sede legale di moltissimi colossi multinazionali. La media europea è comunque del 41 per cento ed anche la media italiana è simile. Questi confronti ci permettono di dire che predicare il no euro o il sì euro è del tutto indifferente, perché le medie, come dati, sono alla pari. L'Italia però ha purtroppo tutti gli indicatori che si collocano verso l'alto;

mi potrà chiedere perché non ho riservato la lettura di questi valori all'intervento sulla manovra di bilancio e li ora. Lei dovrà trattare con Paesi che hanno chiesto a noi i compiti a casa (le famose raccomandazioni della Commissione, periodiche e spesso dettagliate), che in molti casi alcuni di loro hanno svolto, altri, come la Francia, non hanno svolto i risultati si vedono. Ci sono stati Paesi certamente virtuosi, anche perché la loro economia cresce ad un ritmo superiore al nostro e il loro PIL è salito ad un ritmo superiore al nostro. E quindi innanzitutto dobbiamo dare garanzie nel Consiglio europeo che non butteremo via il maggior *deficit*, che non ci spaventa come Gruppo, che abbiamo chiesto come Paese Italia, che questo Governo ha chiesto di poter utilizzare, ma che lo utilizzeremo per fare investimenti.

anche quelle ipotesi di bilancio tracciate nel quadro finanziario pluriennale del *budget* europeo, che non si chiude certamente dopodomani, ma di cui si parlerà

che sono determinanti per la nostra filiera agroalimentare, che è uno dei motori del Paese. Così come dobbiamo negoziare i trasferimenti dei fondi di coesione, di cui il nostro Mezzogiorno - lo dice uno del Nord - ha fortemente bisogno. Nel frattempo, certamente, lo sforzo del Governo e lo sforzo degli italiani è quello di spendere bene, meglio e in modo efficiente i fondi relativi alla programmazione 2014-2021 e alla riprogrammazione che può essere fatta ancora in questi giorni, peraltro con utilità a favore del bilancio dello Stato. Lei ha ricordato anche un altro fenomeno, di cui l'Italia ha dovuto farsi carico senza l'appoggio o con un marginale appoggio dell'Europa: il fenomeno migratorio. Ci associamo a tutto questo; è una questione che non deve essere italiana, ma deve essere europea. Va rammentato purtroppo che il nostro è anche un Paese fragilissimo dal punto di vista idrogeologico. Ahimè, abbiamo tutto il bello, ma anche tutto il brutto, tra cui i terremoti.

abbiamo la TAV, che è un'opera europea, come lo è il tunnel del Brennero. La prima viene costruita verso la Francia e il secondo verso l'Austria:

Bene, questo è frutto di un impegno del passato; la credibilità si mantiene anche mantenendo fede agli impegni, perché gli impegni li ha presi l'Italia, non li ha presi questo o quel Governo. Si tratta di uno dei punti importanti.

non si debba parlare dello zero virgola, ma che sia necessario fornire rassicurazioni al resto d'Europa su un percorso virtuoso che l'Italia deve e può portare avanti, rispettando le regole esistenti, ma con la ferma volontà di cambiarle. Presidente Conte, l'Italia è un Paese fondatore dell'Europa: ha il diritto e il dovere di chiedere la riformulazione di regole che ha condiviso, che potevano valere dieci o venti anni fa e che oggi, con il quadro purtroppo fragile del sistema europeo, devono essere cambiate.

Presidente del Consiglio, rappresentanti del Governo, gentili colleghi, il bilancio pluriennale dell'Unione europea

come è stato anche ricordato in quest'Aula - l'esiguità dei fondi del bilancio, ottenuti in gran parte dai trasferimenti statali. È un bilancio largamente insufficiente per portare avanti misure effettive di crescita economica. Di positivo, tuttavia, ci sono gli interventi a sostegno della sicurezza e della gestione del fenomeno migratorio, oltre che il rafforzamento di quei programmi aventi un valore aggiunto europeo, per noi del MoVimento 5 Stelle molto importante in particolare nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, del clima e dell'ambiente e in favore dei giovani. Una parte significativa è destinata alle relazioni esterne. Grande attenzione va posta, a mio avviso, al prossimo vertice della Lega degli Stati Arabi in programma il 24 e il 25 febbraio del 2019. È l'occasione per un rilancio delle politiche euromediterranee, troppo spesso e frettolosamente abbandonate, riprendendo temi e obiettivi di quella Conferenza di Barcellona del 1995 per la pace e la sicurezza del Mediterraneo e per più stretti rapporti con i Paesi del continente africano. Sulla Brexit, non va trascurato, oltre che un negoziato per un'equa soluzione di questa fuoruscita del Regno Unito dall'Unione europea, un negoziato parallelo il Regno Unito da parte dell'Italia, fondato sulla reciprocità, ricordando che sono 700.000 i cittadini italiani residenti in Regno Unito e che hanno bisogno della massima attenzione da parte del nostro Governo. Sulla ricerca e innovazione ho già avuto modo di intervenire in questa Aula su una importante infrastruttura tecnologica, l'Einstein telescope, un progetto per la misurazione delle onde gravitazionali È un'occasione da non perdere, ma occorre muoversi con decisione e a livello politico perché altri Stati non ci scavalchino. È essenziale, signor Presidente, che il progetto italiano rientri ufficialmente nella *road map* ESFRI, poiché nell'agosto del 2019 verrà scelto quello migliore. L'Europa appare oggi sospesa tra conservazione degli attuali assetti e timidi tentativi di rilancio di un'Europa politica, che possa esprimere una posizione forte per governare i processi della globalizzazione. La visione tedesca, quella di un Europa confederale, fondata su regole di bilancio gestite in termini esclusivamente ragionieristici, che affida agli Stati i compiti da svolgere a casa propria, non può essere l'unica strada. L'Europa deve evolvere in senso federale, ma per questo occorre ripensare criticamente al principio di sussidiarietà, Il principio, come è noto impone, che le decisioni vadano prese, per quanto possibile, al livello più vicino ai cittadini. Da anni stiamo assistendo, invece, ad uno svuotamento dei poteri locali a tutto vantaggio della burocrazia centrale; e i territori si sentono soffocati da scelte calate dall'alto che, di fatto, bloccano le possibilità di crescita. Un esempio è rappresentato dal Comitato europeo delle regioni, organismo che dovrebbe rappresentare idealmente, ma non solo, l'articolazione istituzionale dell'Europa dei popoli ma che è totalmente privo di poteri, condannato ad essere un orpello sostanzialmente inutile. Anche i Parlamenti nazionali hanno un ruolo veramente marginale nella costruzione europea e questo nonostante quanto affermano i protocolli allegati al Trattato di Lisbona. Noi abbiamo assistito recentemente alla bocciatura da parte della Commissione e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (o di gran parte dei Ministri) della nostra legge di bilancio. Ci hanno detto di rifare, ancora una volta, i compiti a casa. Sulla base del principio di sussidiarietà, però, chi deve decidere il bilancio di uno Stato? Quale sia il bene dell'Italia lo sa il Governo che rappresenta il popolo italiano, più che Bruxelles. Sappiamo che essere nell'eurozona comporta vincoli e opportunità, ma ciò non giustifica frasi come quella del Cancelliere austriaco, che riferendosi all'Italia ha dichiarato che l'Austria non è disposta a pagare i debiti di altri Stati. affermazioni del tutto fuori luogo, perché il Governo italiano non chiede affatto che il suo debito venga spalmato tra le altre nazioni dell'Unione europea, ma il sacrosanto diritto di decidere le politiche di crescita economica. Quando si tratta, ad esempio, di considerare problemi importanti per l'economia e la crescita civile di una parte considerevole di europei, come quelli delle grandi e piccole isole, l'Europa non adotta lo stesso rigore formale per verificare se viene rispettata la tutela del principio di insularità. Da un lato si afferma pomposamente le politiche di concorrenza dell'Unione europea garantiscono che le imprese competano in modo leale e in condizioni di parità nel mercato interno europeo. Con il Trattato di Amsterdam si riconosce la tutela delle regioni meno favorite o insulari. L'Unione europea è sempre pronta ad intervenire e a imporre severe prescrizioni in settori che interessano i Paesi forti e continua invece a far finta di niente e a non riconoscere il diritto al riequilibrio delle regioni che essa stessa definisce sfavorite. però il gioco l'abbiamo capito: da un lato nei documenti ufficiali si declamano i succitati principi, dall'altro lato l'Unione europea è fortemente matrigna e fa molti pesi e molte misure. I cittadini che risiedono nelle isole, come il sottoscritto, non chiedono condizioni di favore, ma di riequilibrio: vogliono competere alla pari e questo è un diritto sancito, oltre che dalla nostra Costituzione, dalle norme europee. Signor Presidente del Consiglio, concludo affermando che l'Italia, come è stato ampiamente riconosciuto, è uno dei Paesi fondatori dell'Unione europea ed è da troppo tempo che i nostri *partner* europei ci guardano come un problema e non come una grande risorsa. Negli ultimi anni ci siamo quasi rassegnati a questa condizione, maturando una sorta di complesso di inferiorità. Un grande italiano, Antonio Gramsci, diceva a proposito della sua sardità: «Io sono un sardo senza complessi psicologici». Tale sentimento si adatta bene alla presente realtà italiana nei suoi rapporti con l'Unione europea. Non dobbiamo avere né complessi di inferiorità, né di superiorità, ma vogliamo semplicemente concorrere alla pari dei nostri *partner* europei al benessere nostro e dell'Europa. *(Applausi dai

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate.

del senatore Marcucci. Mi preme inoltre sottolineare la conclusione della COP24, che purtroppo ha avuto un esito molto pesante per quel che riguarda i signori del petrolio, che hanno tentato di di chiudere sul documento conclusivo. Auspichiamo che il nostro Paese ricordi all'Unione europea che siamo i *leader* per quel che riguarda tutti gli interventi strutturali per l'attuazione dell'Accordo di Parigi.

quando ci fu il Consiglio europeo della fine dello scorso giugno, per il quale si era molto preparato, addirittura con due incontri precedenti con il presidente della Repubblica francese Macron, prima a Parigi e poi a Roma. lei era uscito da quel Consiglio europeo felice e trionfalista, dichiarando: «L'Italia non è più sola». Questo disse dopo quel Consiglio europeo: l'Italia non era più sola e non solo con riferimento ai migranti, perché aveva percepito un cambio di paradigma dell'Europa, un cambio di passo. Ebbene, signor Presidente, può dire la stessa cosa oggi? L'Italia non è più sola, come aveva affermato sei mesi fa? Può dire oggi che c'è stato un cambio di paradigma e un cambio di passo in Europa in questi sei mesi? Perché l'Italia oggi è più sola di sei mesi fa? Perché l'Europa non ha cambiato paradigma? Perché - lo chiedo ai colleghi della Lega - i Governi sovranisti europei sono contro l'Italia? Perché il cancelliere austriaco Kurz ha detto quelle parole in riferimento alla manovra economica italiana? Perché la manovra economica italiana, cari colleghi della Lega, non è una manovra sovranista, ma è purtroppo una assistenzialista, che disperde le risorse, punisce le imprese (6,5 miliardi di euro di più tasse per le imprese). La pressione fiscale aumenta nel 2020 e verosimilmente nel 2019. Nel frattempo, anche grazie al decreto-legge dignità, 647 disoccupati in più al giorno; 27 negozi al giorno che chiudono; 5 miliardi di euro di costi in più per lo *spread*, secondo la Banca d'Italia il prossimo anno; 9 miliardi di euro di costi in più nel 2020. L'Italia è più sola perché ha presentato una manovra economica che nemmeno noi conosciamo. Presidente del Consiglio, ieri è iniziata in quest'Aula del Senato la sessione di bilancio. Su quale bilancio? Siamo all'11 dicembre, in procinto dell'esercizio provvisorio. La Camera, per la prima volta nella sua storia, ha votato un bilancio con dei saldi senza conoscere le misure del bilancio, senza conoscere soprattutto le due principali misure su cui vuoi puntate. In primo luogo, il cosiddetto reddito di cittadinanza: abbiamo letto e gli italiani hanno ascoltato credo sette versioni diverse del reddito di cittadinanza. Qual è la carta vera tra le carte false che avete presentato a noi, agli italiani e all'Europa? Quando ce lo direte, a sessione di bilancio finita con il maxiemendamento finale? Quando lo direte all'Europa? Della legge o della riforma della Fornero abbiamo letto nove versioni diverse; l'ultima ieri, secondo cui entrerebbe subito in vigore senza penalizzazione per le pensioni. Quale carta è vera tra le nove che avete annunciato? Le altre otto sono *fake news*.

quale accordo sui rimpatri avete fatto in questi sei mesi? Quanti ne ha fatti l'Europa, che si era impegnata a farli? Quanti? Nessuno. Quante espulsioni sono state fatte in questi sei mesi

Siete inadempienti voi per primi, rispetto agli impegni presi in Europa. Ebbene, è una situazione drammatica perché si discute, per la prima volta in Europa (e vi dovete confrontare), di una

A doverci appellare che far fallire l'Italia è cosa troppo grande per l'Europa? Questo è il grado di contrattazione che siete in condizioni di attuare rispetto a una manovra finanziaria di cui non conosciamo nulla e in cui non c'è nulla per lo sviluppo e per le imprese? Intanto, secondo l'Istat, nel terzo trimestre di quest'anno siamo già a crescita sotto zero e, ove ciò si verificasse anche nel trimestre conclusivo dell'anno i dati sulla produzione industriale sono drammatici), già a gennaio verrebbe certificata la recessione: dopo due trimestri consecutivi a crescita sotto zero, infatti, vi è la recessione. Altro che crescita del prodotto interno lordo all'1,5 per cento quando ancora ieri le maggiori statistiche parlavano di appena lo 0,4 per cento. Si poteva e si doveva andare in Europa a testa alta, con una manovra economica sovranista,

In piazza il *leader* Salvini ha detto che avrebbe trattato lui, è lui che tratterà i buoni mandati con l'Europa, e che il giorno dopo ha ricevuto le imprese; è lui che tratta con le imprese, non il ministro Di Maio o lei: avete ricevuto i sindacati e le imprese mesi, sei mesi in cui non li avete ascoltati e non lo fate ancora oggi con la manovra. Ebbene, mi auguro che sia davvero Salvini a trattare con l'Europa. Mi auguro che sia davvero Salvini a fare i provvedimenti per le imprese; vorrebbe dire che questo Governo è finito e che Salvini fa il Presidente del Consiglio: ci potremmo anche stare, con un programma sovranista, che punti allo sviluppo, sugli investimenti sulle infrastrutture, cioè sulle cose necessarie per creare impresa e lavoro. il programma vuoto, di cartapesta, con le carte false con cui vi presentate in Europa, quale può essere la risposta dell'Europa? Voi condannate non questo Governo, ma l'Italia e i più giovani a una procedura di infrazione sul debito che è un capestro per lo sviluppo del Paese e per le giovani generazioni, esattamente il contrario di quello che raccontate nei *social network* e talvolta anche in quest'Aula. Vi invito a un sussulto di responsabilità: se sarete responsabili, cambiando davvero il senso della manovra, verso lo sviluppo, le infrastrutture, gli investimenti e il lavoro, allora noi ci siamo. Altrimenti, purtroppo, la condanna non dell'Europa - di cui ci importa fino a un certo punto - ma del Paese che sarà in recessione, quella sì, sarà grave e su quella dovrete rendere conto davvero agli italiani. madre del soldato David Tobini, caduto in Afghanistan.

ci rivolgiamo al presidente Conte, nei confronti del quale vi è una comprensione umana, non certo politica, per il compito che lo aspetta; un compito maledettamente complicato, a fronte delle grandi sfide che abbiamo davanti, in un'Europa che sta cambiando, anche nelle sue istituzioni europee. Penso alle sfide dell'unione economica e monetaria, al bilancio europeo e alla alla sfida della Brexit, che spinge tutti noi a chiederci se l'Europa possa andare avanti così. Noi pensiamo che un organismo sovranazionale, originale e straordinario come l'Europa vada coltivato e custodito con la massima attenzione e non messo a rischio con dichiarazioni irresponsabili. Ci sono poi le sfide alle nostre frontiere, le minacce che possono arrivare da Sud e non solo, le relazioni esterne. Quindi, dentro questo mondo complicato lei si trova ad affrontare una sfida da far tremare i polsi, quella cui la sottopongono i suoi due vice nelle dichiarazioni contraddittorie di questi giorni, che fanno diventare il confronto con l'Europa non un confronto vivace, come è fisiologico ci sia, portato avanti anche dai Governi precedenti, ma un confronto che può assumere, se portato alle estreme conseguenze, toni drammatici. Non si scherza sul debito che abbiamo

In passato, Governi che si rendevano conto della difficoltà della sfida provavano a lanciare dei messaggi alle altre forze di opposizione per andare avanti con un mandato molto ampio

e, quindi, se fa una brutta figura l'Italia la fa tutto il Paese, noi compresi che siamo all'opposizione. Lo dico perché sulla parte del bilancio europeo vediamo indubbiamente dei passi avanti, soprattutto dal punto di vista delle politiche regionali, dove aumentano i miliardi che saranno a disposizione del nostro territorio, delle aree metropolitane del nostro Paese. Così non è sulla sull'agricoltura; non sappiamo se ci sono dei margini. Probabilmente quando ci sarà la revisione a metà mandato sarà uno dei temi su cui lavorare. L'Italia avrà 4 miliardi di euro in meno e sarà problematico da quel punto di vista rispondere anche agli interessi dei nostri territori, dei nostri operatori e di chi lavora nel campo dell'agricoltura. Lo dico perché ci sono dei risultati positivi, ma altri da cogliere. Anche sulle sfide sull'Unione economica e monetaria sono stati fatti passi in avanti importanti, che sono dentro la storia del nostro Paese. Il lavoro fatto dai Governi precedenti viene a maturazione. Penso al fondo per la risoluzione delle crisi bancarie e all'attenzione nei confronti dei nostri risparmiatori

dei Paesi che fanno parte dell'Euro. Serve di più; serve anche un meccanismo di stabilizzazione, un'assicurazione sui depositi e qui servono le alleanze. alleanze. Sul versante dei fondi per l'agricoltura, per esempio, un asse con la Francia sarebbe fondamentale. C'è bisogno di un recupero delle relazioni diplomatiche positive, nei confronti della Francia, dei nostri alleati storici, con una diminuzione di un confronto

di un grande successo che lei stesso ha portato in quest'Aula parlando delle piattaforme regionali per riconoscere subito chi è migrante economico e chi è rifugiato di tutto ciò non ne troviamo più traccia. Nessuna notizia neanche sui centri nei Paesi membri

Noi precedentemente avevamo affermato il principio secondo cui la redistribuzione dei rifugiati dovesse essere obbligatoria. Ebbene, questo principio è saltato e si è passati dalla redistribuzione obbligatoria alla redistribuzione su base volontaria; quindi, un arretramento rispetto al passato. Sul versante delle politiche legate all'asilo dei rifugiati il trattato dell'Unione europea parla chiaro: è una di quelle materie su cui si può decidere a maggioranza. Noi abbiamo accettato che su un tema delicato come Dublino si decida all'unanimità; quindi, anche in questo caso un passo indietro dovuto alle alleanze che abbiamo scelto. Abbiamo deciso di allearci e di avere un rapporto privilegiato con i Paesi di Visegrád e questo che conta, sui temi principali i Paesi di Visegrád si voltano dall'altra parte, tanto che sono stati i primi - loro, insieme all'Austria - a dire che non accettavano deroghe alla normativa europea e che alla fine la manovra avrebbe dovuto rispettare le stesse regole che valgono per gli altri Paesi europei. Da questo punto di vista, di vista, una profonda riflessione sulle scelte che avete fatto rispetto alla costruzione delle alleanze - che sono fondamentali nel gioco europeo per portare a casa i risultati - deve essere fatta, ed è il motivo per cui voteremo evidentemente contro la risoluzione della maggioranza. il Global compact for migration abbiamo fatto una grandissima figuraccia, Presidente. Il 26 settembre l'Assemblea delle Nazioni Unite ha detto di andare avanti sul Global compact perché non era uno strumento vincolante, ma un quadro di collaborazione positivo tra Paesi che riconoscevano un punto fondamentale su cui non si può transigere, ovvero il rispetto dei diritti umani: salvare vite e allo stesso tempo collaborare per infliggere un duro colpo ai trafficanti di esseri umani. Questo dice il Global compact e noi abbiamo deciso di accettarlo; era giusto.

Si tratta di un passo indietro per il lavoro che abbiamo sempre fatto in Europa, dove siamo stati il Paese guida da questo punto di vista. Rispetto alla Libia, non siamo riusciti ad averla per

non bastano le parole che ha detto: serve una condanna molto chiara. Pensiamo che le sanzioni servano e sono uno strumento per dire alla Russia che non può fare quello che vuole:

l'idea delle piccole patrie ha portato all'unico vero, grande conflitto nella terra europea negli anni Novanta. Su questi temi non possiamo scherzare; ci sono certamente da valutazioni dal punto di vista economico, ma non possiamo venire meno ai nostri valori e ai principi fondamentali su cui si basano l'Europa e i Paesi democratici. Da ultimo - e concludo, Presidente

la richiesta di inserire la lotta contro l'antisemitismo. Penso che questo sarebbe un segnale importante e forte, all'indomani dell'ultimo atto che abbiamo visto proprio ieri, quando sono state rimosse le venti «pietre d'inciampo» nel Rione Monti. Ebbene, serve una risposta chiara anche a livello europeo per cui, senza se e senza ma, senza infingimenti, senza senza dare sponda a episodi di intolleranza e di razzismo, come Europa si possa esprimere una posizione forte e chiara contro ogni razzismo, contro ogni forma di xenofobia e in una lotta senza se e senza ma agli episodi legati all'antisemitismo.

l'avvocato difensore del popolo italiano, delle parole che non mi parvero ovvie. Non lo erano affatto, per chi come me per tanto tempo non si era sentito rappresentato e difeso dalla classe dirigente di questo Paese, forse anche per quell'atteggiamento che abbiamo sentito echeggiare in alcuni interventi di chi mi ha preceduto, per questa volontà di mostrare sempre che l'Italia era avanti su certe agende, quasi dovesse scusarsi di un complesso di inferiorità che, sinceramente, alla prova dei fatti, come anche documenterò, non mi sembrava fondato. Per la prima volta sentivo un politico esprimere, con parole sincere, il desiderio di difendere gli interessi del Paese. Mi sento in colpa, quindi, perché dovrò rispondere a queste parole non ovvie con un paio di ovvietà. La prima ovvietà, cominciando dalla fine, è che naturalmente io, parlamentare di maggioranza, esprimerò un voto favorevole alla risoluzione presentata dalla maggioranza. È una cosa ovvia, come è ovvio che dalle opposizioni lei abbia avuto delle critiche (diciamolo pure, senza sminuirne il valore: le solite critiche). Ci sono cose anche più ovvie di questa, che però stranamente fanno notizia in questi giorni. È assolutamente ovvio, ad esempio, perlomeno a me - non vorrei sembrare supponente che in questo momento stiano esplodendo nel Nord della meravigliosa famiglia europea le profonde contraddizioni del progetto così come è stato concepito. Non mi riferisco semplicemente alla manifestazione più variopinta e più sgargiante, quella dei *gilet* gialli, che già hanno piegato il Governo di Macron, la grande speranza degli schieramenti progressisti europei, ma mi riferisco anche a un grafico che qualcuno di voi avrà visto, quello che sovrappone l'andamento delle azioni di Deutsche Bank all'andamento delle azioni di Lehman Brothers prima dei noti fatti che la colpirono. L'andamento è assolutamente speculare e sovrapponibile, il che non lascia presagire nulla di buono sul fronte occidentale, quello francese, in termini sociali e nulla di buono sul fronte orientale, quello tedesco, in termini bancari. Non lo dico per *Schadenfreude*, che è la parola che noi europei utilizziamo per indicare la gioia vigliacca di chi si compiace delle sciagure che accadono all'avversario (parola che casualmente è una parola tedesca). Lo dico per fare una riflessione diversa: è del tutto evidente che stanno cambiando i rapporti di forza in Europa e quindi lei, come avvocato difensore del popolo italiano, almeno in linea teorica dovrebbe avere la strada spianata. Questo però richiede attenzione. Il momento è delicato e sono stato particolarmente colpito e rassicurato dal fatto di vedere che lei è consapevole della delicatezza del momento e del fatto che il bilancio dell'Unione europea è un documento che ci impegna per sette anni e quindi è molto importante riflettere su quanto sia opportuno valutarlo in una situazione nella quale gli assetti politici congelati nelle istituzioni europee sono totalmente scollati da quelli che la società europea e gli elettori europei stanno esprimendo pressoché ovunque. La Francia, per uscire dalla situazione delicata nella quale si trova, ha annunciato che farà la cosa più ovvia, quella che si deve fare quando c'è una situazione recessiva: farà una politica espansiva.

meno augusta di questa, una sede televisiva, di fronte a uno dei competenti (di quelli che sanno tutto e che quindi non hanno fatto molto), ovvero che potrebbe anche superare il 4 per cento. In questo scenario, noi stiamo parlando di un -0,2 per cento per il nostro Paese, che quindi appare chiaramente

perché si vedrebbe che argomenti pseudoeconomici vengono utilizzati come strumento di pressione e direi quasi di bullismo politico. A noi viene detto che però la Francia può permetterselo perché ha poco debito. È È vero, l'Italia ha un grande debito, che è aumentato durante la crisi, nonostante noi fossimo governati dai sacerdoti dell'*austerity*, alcuni dei quali siedono anche in questo consesso. il debito italiano è aumentato di 686 miliardi di euro e sto parlando dell'incremento dal 2007 al 2018; nello stesso periodo quello francese è aumentato di 1.025 miliardi di euro, cioè più di 300 miliardi in più. se vogliamo parlare di quella spesa che ci viene dipinta come fuori controllo, il flusso della spesa corrente complessiva del Governo italiano nello stesso periodo è aumentato di 95 miliardi di euro

una produttività e redditi che languono, è semplicemente per un motivo banale: finora i nostri Governi non hanno avuto il coraggio di fare quello che - grazie a Dio - l'Esecutivo che noi come maggioranza sosteniamo ha avuto il coraggio di realizzare, cioè politiche anticicliche. Inoltre, visto che lei ha espresso l'urgenza di un cambiamento, va detto che dovrebbe trattarsi anche di un cambiamento delle regole, perché per chi voglia entrare nel dettaglio delle regole europee è importante sapere che quando una crisi malgestita lascia una cicatrice nella crescita di un Paese, secondo le regole europee Paese si condanna a smettere di crescere, per il semplice motivo che il cosiddetto PIL potenziale è una misura che non guarda allo stato oggettivo dell'economia ma alla storia passata, incorpora tutti gli *shock* negativi. Pertanto, adesso per l'Europa è normale che l'Italia sia un Paese con la disoccupazione all'11 per cento e noi questo non possiamo tollerarlo e non possiamo permettercelo. - e concludo, Presidente ne ha rimarcato l'importanza dicendo che è un bene da tutelare al pari di quella fine quella finanziaria; stabilità finanziaria che neanche la Commissione europea, non esattamente benevola con noi per motivi che non capiamo sinceramente e che ci amareggiano, è riuscita a dimostrare venga infranta da questa manovra; ebbene, quando voi per primi parlavate della stabilità sociale come bene da tutelare, io vedevo dei sorrisetti di circostanza, come se quella fosse una scusa. Quello che sta succedendo in Francia invece ci dimostra che avevate ragione voi *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)* e che se in Italia riusciremo ad evitare scenari di questo tipo, sarà perché abbiamo avuto un Governo proattivo nel difendere questo bene, nel difendere la civile convivenza dei cittadini. Pertanto - mi ripeto - per questo motivo

gli auguri con tutta sincerità; il Gruppo Forza Italia le augura di poter difendere con successo e con efficacia le ragioni e gli interessi degli italiani nel prossimo Consiglio europeo.

al Governo come all'opposizione, perché nell'Unione europea passi una linea espansiva che non penalizzi Paesi come l'Italia, che si trovano gravati di un debito pubblico accumulato nei decenni precedenti.

adesso le tocca trattare e tirare molto meno che dritto (non so se storto, ma quanto meno un po' indietro). Sul tema dell'immigrazione è difficile che gli altri Paesi ci ascoltino visto che siamo isolati e ci troviamo in una situazione molto particolare. La collocazione geografica dell'Itala

Perché lo facciamo? Ho l'impressione che la ragione sia che ce lo chiede l'Europa. Questa è una vecchia e criticatissima frase che viene attribuita sempre agli avversari, ma adesso (anche la scorsa settimana, su sfalci e potature, argomento assai terra terra rispetto ai massimi sistemi europei) abbiamo avuto la stessa risposta: votiamo una norma assurda perché ce lo chiede l'Europa. Cosa è cambiato? Oltre a dover seguire molte delle indicazioni europee anche quando non siamo d'accordo,

che parlasse di tempi al presente o di quello che avviene domani, non certo che dopo quaranta giorni di legge di bilancio alla Camera e quando siamo ormai a dieci giorni da quando il Senato dovrebbe chiudere la discussione, ancora non sappiamo nulla. La Commissione bilancio discute, è lì e lavora lodevolmente, ma non avendo l'emendamento evidentemente promesso dal

che le lettere dell'Unione europea fossero dette così per dire e che essa non facesse sul serio, si è scoperto poi che non facevano sul serio gli esponenti italiani, che dicevano «non cambieremo di un millimetro». Su che cosa sta trattando? Lei ci chiede un mandato in bianco che la sua maggioranza le darà, ma noi non le daremo un mandato in bianco. Sappia però che se lei saprà mettere gli interessi dell'Italia al di sopra degli interessi dei singoli partiti della maggioranza e della coalizione del contratto di Governo, lei avrà il nostro sostegno. Certo, non ha un compito facile; ottenere qualcosa dall'Unione europea che si attacca ogni giorno, è davvero un compito difficile, ma se lei lo facesse, noi la sosterremmo, perché per Forza Italia vengono prima gli interessi degli italiani, sia che siamo al Governo sia che siamo all'opposizione.

da componente della Commissione politiche dell'Unione europea sono onorata di prendere la parola per la prima volta in questa prestigiosa Assemblea, al cospetto del nostro Presidente del Consiglio. La sagge parole del presidente Conte ci hanno fatto capire che l'Italia, grazie al Governo del cambiamento, sta cominciando a giocare un ruolo da protagonista; il ruolo che le spetta per storia, prestigio e peso culturale. Per la prima volta dopo tanti anni non andiamo più in Europa a discutere, elemosinando concessioni con il capo cosparso di cenere, ma a testa alta come interlocutori credibili in grado di affrontare da pari a pari le varie tematiche che si presentano sul tavolo della mediazione politica e lo facciamo perché crediamo ancora in un'Europa espressione di democrazia, pluralismo e rispetto delle differenze, che funga da sintesi rispetto alle decisioni dei Parlamenti nazionali. Oggi siamo qui a discutere questa importante risoluzione; un impegno complesso, composito, uno di quei passi indispensabili volti a costruire l'identità dell'Europa. In questo quadro comunitario si rende necessario il perseguimento della strategia per il mercato unico digitale, che sarà certamente cruciale per stimolare la competitività, l'innovazione e la sostenibilità dell'economia nazionale e di quella europea. Secondo la Commissione europea un mercato unico digitale pienamente funzionante potrebbe apportare fino a 415 miliardi di euro annui all'economia dell'Unione europea e permetterle di diventare un *leader* digitale a livello globale. La realizzazione a livello europeo di politiche di contrasto della delocalizzazione fiscale delle imprese nei Paesi extra Unione europea, soprattutto con riferimento alle grandi società multinazionali che operano nel mercato digitale, appare oggi più che mai necessaria per ottenere una redistribuzione degli ingenti profitti realizzati da queste realtà internazionali e un contestuale rafforzamento della domanda aggregata. In tema di immigrazione troviamo imprescindibile avviare iniziative europee per intensificare il contrasto alle reti dei trafficanti di persone e rafforzare ulteriormente la cooperazione con i Paesi terzi in materia di indagine, arresto e perseguimento di soggetti dediti al traffico e alla tratta di esseri umani. Prioritaria risulta inoltre l'adozione immediata e condivisa a livello degli Stati membri dell'Unione europea di una strategia europea strutturata su politiche comuni nell'immigrazione, con una condivisione delle responsabilità e un'equa ripartizione delle pressioni derivanti dai flussi migratori, in particolare dei salvati in mare, garantendo l'impiego delle risorse nel modo più efficiente possibile ed elaborando norme comuni per la sorveglianza delle frontiere esterne, la cui difesa deve essere necessariamente condivisa dagli Stati membri. Signor Presidente del Consiglio, questa risoluzione ci spinge ad un'analisi rispetto alla quale non possiamo rimanere indifferenti e che l'onestà intellettuale ci impone. Oramai tutti noi, anche da posizioni diametralmente opposte, abbiamo consolidato negli ultimi tempi una consapevolezza diffusa, che questa Europa, così come è, non funziona e va cambiata con intelligenza e sacrificio. L'Unione che abbiamo conosciuto in quest'ultimo decennio ha fallito la *mission* che era chiamata a realizzare, cioè creare i cittadini europei e avvicinarli alle istituzioni che li rappresentano. Questo dato di fatto richiede una serie di interventi da porre sul tavolo delle trattative che guideranno la sua mediazione con l'Unione europea sulla nostra manovra di stabilità. Siamo certi che, grazie alle sue grandi qualità di mediatore, riuscirà nell'impresa. Un coordinamento efficiente delle politiche fiscali nazionali per garantire l'efficacia della politica monetaria comune è reso necessario dalla stretta dipendenza intercorrente tra bilancio pubblico e stabilità monetaria, bancaria e finanziaria. Solo una combinazione coerente ed efficace di politica dell'offerta e della domanda aggregata, generatrice di moltiplicatori economici, può evitare che l'economia europea e la stessa stabilità monetaria comune ristagni ed entri in un tunnel involutivo dal quale sarà impossibile uscire. Si rende quindi indispensabile una ridefinizione della politica fiscale europea che sia coerente con quella dei singoli Stati. La via maestra passa attraverso il completamento dell'Unione politica e la ristrutturazione dell'architettura istituzionale dell'Unione. C'è da dire che questo Governo si sta assumendo anche le responsabilità derivanti dagli impegni scellerati assunti dai Governi precedenti; ma non si sta certamente tirando indietro. Oggi è imperativo agire con decisione per rilanciare le nostre economie e contrastare la disoccupazione e il dilagare della povertà. Per questo motivo noi del MoVimento 5 Stelle dobbiamo insistere sulla via del dialogo con la Commissione. La strada maestra non può che essere quella indicata dal Presidente della Repubblica nel corso della sua recente visita in Svezia: dialogare e recuperare *l'esprit d'Europe*. L'Italia vuole dialogare. Sta agli altri dimostrare di volersi occupare seriamente del futuro dell'Unione europea, senza arroccarsi su posizioni indifendibili e insostenibili da ogni punto di vista. Desideriamo dare espressione alla speciale comunità di tradizioni e sensibilità che sono proprie dei popoli europei. Vogliamo arricchire la solidarietà atlantica facendo sì che in essa si inserisca l'Europa con una voce propria, con le caratteristiche connaturate alla propria civiltà, con le sue particolari esigenze e attitudini. Lo sguardo va posto all'Europa dopo l'Europa, alla necessità di sotterrare l'ascia di guerra, che le forze nazionali possono brandire in maniera autodistruttiva, e di creare le basi per una nuova alleanza trasversale tra popoli e classi, nella ricerca di interessi comuni, riprogettando gli organi di rappresentanza dell'Unione e legittimandone l'esistenza. L'Unione europea deve riaffermare la propria identità e lo deve fare ora, senza ulteriori rinvii, perché nuove sfide attendono dietro l'angolo, a partire dalle biotecnologie e dall'intelligenza artificiale. L'Europa è chiamata a rispondere alla sfida lanciata da colossi come Cina e Stati Uniti anche sul piano della sovranità digitale, attraverso significative riforme fiscali intese a favorire l'insediamento di nuovi poli cibernetici e a frenare la fuga di cervelli. Chi meglio dell'Italia potrebbe candidarsi a ospitare una Silicon Valley europea? Dato che questa Unione europea non ha risolto tutti i suoi difetti costitutivi e non ha affrontato le criticità vitali per la sua stessa sussistenza, non instilla e non infonde grande fiducia nei suoi veri azionisti, che sono i 500 milioni di abitanti che la popolano, per quale motivo dovremmo avere così paura del cambiamento? Perché dovremmo pensare che ridisegnare nuove regole basate non più su *austerity* e politiche restrittive, ma sul sostegno alla domanda, debba condurci verso il baratro? Per quale motivo non dovremmo adottare una prospettiva diversa da quella che ci ha portato ad addentrarci in questa buia crisi identitaria, da cui non sappiamo uscire? Spesso l'evoluzione sociale è passata attraverso una modifica delle condizioni socio-economiche precostituite e dei convincimenti ideologici dominanti preconfezionati. Continuare a procedere lungo la strada fin qui seguita non ha prodotto miglioramenti; questo è l'unico dato certo. Seguendo questa linea di pensiero, la logica non può che spingerci a cambiare il percorso, per seguirne uno alternativo nella direzione auspicata da questo Governo. Vogliamo un'Europa diversa e innovata; vogliamo che l'Europa torni in mano ai suoi popoli e alle sue nazioni. Vogliamo l'Europa sognata dai suoi ideatori e fondatori: l'Europa di Schuman, di Monnet, di Altiero Spinelli, di Adenauer e De Gasperi; non l'Europa delle aride equazioni normative, degli algoritmi monetari e dell'egemonia tirannica della *troika*. È quella l'Europa che ci piace. È quella l'Europa che ci rinvigorisce l'animo e che ci dà speranza; quell'Europa che, una volta girata pagina, sono sicura lancerà una nuova sfida al mondo, una sfida di cultura, di civiltà, di diritti, di democrazia, di benessere e di solidità economica. Da qui dobbiamo ripartire per sentirci tutti più e meglio europei. Per questi motivi, a nome dell'intero Gruppo MoVimento 5 Stelle, non posso che rinnovare al nostro Presidente del Consiglio il nostro massimo sostegno e la nostra massima stima e considerazione, dichiarando con orgoglio il nostro voto favorevole.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

La Conferenza dei Capigruppo ha rimodulato la trattazione degli argomenti previsti dal calendario della settimana corrente, alla luce dell'anticipazione alla seduta odierna delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo

fino alla sua conclusione e, ove conclusa dalla Commissione, la ratifica della Convenzione di Faro sul patrimonio culturale. Su richiesta di un Gruppo parlamentare, la seduta di domani sarà sospesa tra le ore 12 e le ore 15. L'eventuale seduta già prevista per venerdì 14 non avrà luogo. In relazione alla sessione di bilancio, il termine per la presentazione dei rapporti delle Commissioni alla Commissione bilancio è posticipato alle ore 19 Grazie a tutti relative alla costituzione delle Commissioni bicamerali semplificazione, vigilanza anagrafe tributaria, questioni regionali e controllo enti gestori - annunciate all'Assemblea nella seduta del 4 dicembre scorso - non avranno luogo.

intervengo per segnalare un grave fatto avvenuto questa notte a Roma. Mi riferisco all'incendio che si è sviluppato all'interno dell'impianto dell'AMA sulla Salaria. Questo episodio ha dimostrato per l'ennesima volta che, purtroppo, a Roma i cittadini non si sentono sicuri al di fuori delle loro case.

notevoli problematiche a tutta la popolazione del comprensorio. Vorrei sottolineare che questo episodio poteva essere evitato, anche perché stiamo parlando di un impianto che stava trattando 3.000 tonnellate, quando invece sappiamo che ne potrebbe trattare 600. Tutto ciò, tra l'altro, è aggravato anche dal fatto che esso è sprovvisto di una piazzola dove i camion possano fare manovra:

nessuno aveva dato mai peso a queste situazioni. Vorrei anche far presente che vicino a questi impianti ci sono dei campi agricoli e, anche se oggi è stata

che sicuramente sono nocivi per la salute e, soprattutto, i prodotti che sono stati venduti prima di questo evento.

questo è il momento di dare risposte concrete ai romani, che già un mese fa avevano dimostrato in piazza la contrarietà all'amministrazione e l'amministrazione si era rivelata sorda a queste proteste.

e non vorrei sparare sulla Croce rossa, ma la dignità umana viene persino prima della salute. Come diceva il collega intervenuto prima di me, oggi è scoppiato un incendio a un impianto di rifiuti, il TMB Salario. Ero lì stamattina e c'era una puzza incredibile, una nube nera che ha attraversato il cielo di Roma.

siamo dovuti stare attenti alle previsioni del tempo, per capire dove andava la nuvola e quale nocività avrebbe creato

che raccoglie indifferenziato. L'11 ottobre io stessa, personalmente, ero intervenuto in Assemblea per farmi portavoce delle istanze della popolazione e della richiesta di chiusura di quell'impianto. Il 12 giugno avevamo presentato l'interrogazione parlamentare il 14 novembre il mio collega Andrea Ferrazzi l'ha sollecitata in Commissione ecomafie. E non si sono trovate soluzioni: è questo il problema. Noi dovremmo solo chiedere scusa scusa ai cittadini romani per questo, per non aver trovato soluzioni. C'è stata una recente indagine dell'ARPA Lazio che ha messo nero su bianco quali erano le problematiche di quell'impianto. Il primo cittadino del municipio Giovanni Caudo ho chiesto l'unità di crisi, già da qualche mese, tra Comune, Regione e Ministero. Non vorrei fare una polemica di colore politico, anche se sarebbe facile, perché questa amministrazione è da due anni e mezzo che governa. Però una cosa voglio dirla: non può venire da alti esponenti di

domani saranno sette mesi dalla nostra interrogazione e il ministro Costa non è venuto in Parlamento per riferire su questa situazione. Chiediamo con forza la presenza del ministro Costa perché lui possa riferire, a questo punto anche su una situazione di emergenza della città di Roma e per trovare delle soluzioni. Noi siamo tutti rappresentanti dei cittadini e delle cittadine, qualche forza politica ama dire «portavoce», ma il Parlamento è il luogo nel quale il ministro Costa deve riferire e deve, insieme a noi, trovare soluzioni per ristabilire una vita dignitosa

Vicenda che registra nelle ultime ore nuovi, inquietanti sviluppi: ci sono notizie sulla sottoposizione ad indagine del tesoriere nazionale della Lega Giulio Centemero; ci sono notizie riguardo a perquisizioni avvenute in studi di commercialisti legati al partito del Ministro dell'interno. Nelle settimane e nei mesi scorsi ci sono state altre due novità rispetto all'ultima volta in cui quest'Assemblea si è occupata della vicenda dei 49 milioni oggetto della truffa. È intervenuta la condanna di appello (ormai manca soltanto il terzo grado di giudizio), che ha confermato la colpevolezza degli onorevoli Bossi e Belsito rispetto a questa gravissima mancanza, che ha suscitato profonda inquietudine in tutta l'opinione pubblica. Infine, la vicenda, che ha suscitato polemiche non lievi, della decisione di accordare una rateizzazione in settantasei anni della cifra di 49 milioni che lo Stato deve avere indietro e che il partito del ministro dell'interno Salvini dovrebbe avvertire la necessità di restituire senza indugio per fare un atto di giustizia e compiere un dovere nei confronti dello Stato e degli italiani. Noi vediamo che molte cose cambiano; l'unica cosa che non cambia, l'unica novità che non si registra è l'atteggiamento del Ministro dell'interno, che minimizza, ridimensiona, nega l'evidenza, cerca di mettere la polvere sotto il tappeto. Non riteniamo questo atteggiamento accettabile e per questo annunciamo che nella prima Conferenza dei Capigruppo in cui sarà possibile il Partito Democratico chiederà che il ministro della giustizia Bonafede venga a riferire in Aula sugli sviluppi di questa vicenda. Non è più possibile per nessuno, tantomeno per il Ministro della giustizia fare finta di niente; non lo è nemmeno per il Ministro della giustizia, anzi direi soprattutto per il Ministro della giustizia, dopo quello che abbiamo sentito oggi, ossia le dichiarazioni prima dei due Capigruppo del MoVimento 5 Stelle alla Camera e al Senato, d'Uva e Patuanelli, e poi del vice *premier* Di Maio, i quali hanno detto di essere sicuri che ci sarà trasparenza, di voler trasparenza, che sono certi che il ministro dell'interno Salvini non minimizzerà e darà chiarimenti. Il posto dove i chiarimenti debbono e possono essere meglio dati è il Senato della Repubblica, che tante volte ha discusso di tale questione. Qualche malalingua dice che gli esponenti del MoVimento 5 Stelle adesso chiedono trasparenza e si dicono certi che Salvini non minimizzerà perché voglio allontanare l'attenzione dalle disavventure giudiziarie della famiglia del vice *premier* Di Maio per riportarla sulle disavventure giudiziarie dell'altro Vice *Premier*. Noi non siamo interessati alla dietrologia e ai retroscena. Quando qualcuno chiede trasparenza su fatti così gravi siamo sempre d'accordo. Siamo stati la prima voce che ha chiesto trasparenza e chiarimenti in Parlamento e spesso siamo stati inascoltati. Vogliamo che il Ministro della giustizia venga in Assemblea e siamo sicuri che questa richiesta, se c'è un minimo di senso dello Stato e delle istituzioni, sarà accolta, perché questo è un dovere nei confronti del popolo italiano.

Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 dicembre, una trentina di persone ha occupato abusivamente la casa cantoniera di Oulx, al fine di dare assistenza ai migranti diretti in Francia. Dalla loro pagina Facebook pubblicizzano alla nascita del rifugio autogestito contro le frontiere, contro il decreto Salvini e a favore di coloro che non hanno il pezzo di carta giusto. Sostengono che, da quando il rifugio di Claviere è stato chiuso, sono aumentati gli smarrimenti di migranti e i decessi. Questo è vero, ma non è dovuto alla mancanza di assistenza, bensì è conseguenza della stagione fredda, della neve e delle temperature rigide. Partiamo dal presupposto che, se pur realizzata in un'ottica benevola, dal loro punto di vista, questa postazione non fa altro che aumentare le potenziali vittime della montagna e del gelo, perché illude queste persone di poter attraversare il confine senza troppe difficoltà, incoraggiandole, a meno che la premiata organizzazione del rifugio non fornisca anche la dotazione di *passeur* per favorire l'attraversamento della frontiera. A tal proposito, sottolineo come l'ospitalità e l'accompagnamento in Francia fornito dall'ormai chiuso sottochiesa di Claviere fosse a pagamento. Considerato che gli occupanti, riconducibili ai centri sociali, hanno invaso dei locali abusivamente, forzando serrature e violando una proprietà privata, preso atto, dalle loro parole, che questo atteggiamento è l'ennesimo atto ostile nei confronti dello Stato, accertato che in passato questi benefattori si facevano pagare dagli stessi migranti per le prestazioni fornite e tenuto conto che il loro comportamento non fa altro che incentivare la fuga dai centri dei migranti irregolari, tirandoli fuori dai circuiti dell'assistenza statale e facendo perdere loro ogni diritto, lasciandoli in preda all'illegalità, auspico che lo sgombero della casa cantoniera avvenga al più presto, al fine di riportare la serenità a Oulx e la tranquillità in Valsusa e di garantire l'incolumità dei migranti stessi, ripristinando al tempo stesso la legalità.

motore di tutta la produzione italiana di olio di qualità pregiata. Nello specifico, voglio ricordare i danni che lo scorso febbraio-marzo hanno colpito i territori pugliesi, determinando con le gelate la perdita della quasi totalità delle olive, con conseguenti enormi danni per tutto il settore. Sono molto preoccupata, poiché in questo momento storico la Puglia, già pregiudicata dalla *xylella*, non può permettersi un danno del genere. Per cui chiedo, al di là di ogni specifica responsabilità, di intervenire a sostegno del comparto olivicolo pugliese, eccellenza di tutta l'Italia.

voglio intervenire in Assemblea per ricordare - mi sembra giusto e doveroso - la strage che si è verificata qualche giorno fa nella discoteca «Lanterna Azzurra» di Corinaldo, in provincia di Ancona, che ha gettato nel più profondo sconforto ognuno di noi. Ci sono sei vittime, cinque minorenni, una mamma, settanta feriti, una situazione veramente terribile. Uno sconforto che, tuttavia, ci obbliga a un'attenta e seria La magistratura certamente sta indagando e sta facendo il proprio dovere. Cercherà i responsabili, coloro che hanno provocato questa strage o che hanno concorso a provocare questa strage, ma la politica, secondo me, si deve interrogare su una società che è in *overdose* di diritti e svuotata di doveri, una società che ha messo alla porta i valori più forti e più profondi e ha reciso i legami - se vogliamo trovare una responsabilità di carattere culturale - con la società tradizionale. Dobbiamo anche dirci che in Italia l'attività di controllo sulla sicurezza degli eventi di intrattenimento, soprattutto ai quali partecipano i minori, è assolutamente insufficiente. Occorrono, dunque, più controlli e restrizioni, soprattutto quando di mezzo ci sono dei ragazzi e degli adolescenti. Quali misure applicare? Sarebbe opportuno che il Parlamento e la nostra Aula se ne occupassero con un provvedimento condiviso.

dall'obbligo di apertura e chiusura dei locali in orari diversi rispetto al fatto che partecipino minori oppure persone che minorenni non sono e la chiusura immediata e la revoca della licenza per chi supera il numero di ingressi legalmente consentiti. revoca definitiva per chi ospita individui che vendono o cedono a qualsiasi titolo a minori alcol, fumo e sostanze stupefacenti. Nel nostro ordinamento c'è un articolo poco frequentato e che poco piace a qualcuno e, in particolar modo, alle procure della Repubblica Italiana. È l'articolo n. 309 del 1990. Presidente, l'articolo riguarda l'agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno dei locali.

l'obbligo morale di controllare che nessuno speculi sulla pelle dei nostri ragazzi. Signor Presidente, intervengo anche io sulla questione e, purtroppo, sulle cronache relative al TMB Salario, all'incendio, per chiarire una cosa. Questo evento così importante e dannoso per tutta la città non può essere consegnato alla speculazione politica; questo non può essere consentito a nessuno. Questo incendio danneggia tutti i cittadini romani romani e ritengo, quindi, inopportune le critiche che sono state portate al sindaco Virginia Raggi, che è vittima in rappresentanza dei cittadini romani di questo atto. Sicuramente la procura stabilirà nel prosieguo delle indagini le responsabilità, ma non è un caso che in Italia scoppino almeno 300 roghi che riguardino i rifiuti e non è un caso che il sistema dei rifiuti - è stato provato - è in mano in parecchie Regioni del nostro Paese alla criminalità. Quindi, quanto ha fatto il sindaco Virginia Raggi finora è smontare pezzo per pezzo tutto questo sistema criminale e, se c'è qualcosa di veramente indegno in questo momento in cui dovrebbe esserci una preoccupazione per la salute, è fare speculazioni politiche. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Il ministro Costa ha già parlato con la ASL e con l'ARPA. Non ci sono emergenze, ma è un fatto concreto, ad esempio, che il decreto sicurezza, all'articolo 26, abbia già previsto cosa bisogna fare in questi casi. Finora non c'era stata una normativa che dicesse cosa bisognasse fare in questi momenti. momenti. Adesso bisogna lasciare che le persone impegnate, le autorità e le istituzioni risolvano il problema e lasciare da parte le speculazioni politiche che non interessano né i cittadini né tutti coloro i quali sperano che le cose vengono risolte.

Grazie a tutti